di amministrazione. Anche questa mattina tutta la maggioranza non si è presentata in Commissione (non è la prima volta che accade), impedendo così sostanzialmente il funzionamento della Commissione stessa. Non mi riferisco soltanto alla parte relativa alla nomina del Presidente, per la quale evidentemente assistiamo a uno stallo all'interno delle forze della maggioranza, ma al funzionamento integrale della Commissione, perché non è stato possibile programmare le audizioni, né discutere sullo svolgimento degli ulteriori lavori.

i lavori e tutto ciò che va organizzato in Rai in questo momento è fermo. Volevo lasciarlo agli atti della seduta di oggi, perché ritengo che questa condotta e questa scelta da parte della maggioranza vadano sicuramente stigmatizzate.

in questi mesi purtroppo si sta ripetendo: non siamo in grado, in Commissione di vigilanza Rai, di discutere e di votare sulla Presidenza della Rai. Presidente, la Rai fa parte della storia di questo Paese, ha avuto una grande funzione informativa, formativa e di spettacolo, con livelli altissimi.

di Mediaset, La7 e Sky. La sera e la giornata delle elezioni di quest'ultima tornata elettorale regionale, se i cittadini e le cittadine volevano avere qualche notizia, dovevano andare su queste televisioni *(Applausi)*, perché la Rai non ha dedicato alcun momento di approfondimento e di informazione, anche rispetto a una partita elettorale assolutamente significativa. Moltissimi grandi protagonisti della Rai sono andati in altre televisioni. Allora, Presidente, questo atteggiamento per cui la Presidenza non si concorda e non si discute, non si trovano percorsi che tengano assieme, ma, siccome non si hanno i numeri, si disertano la Commissione di vigilanza e le votazioni, deve finire perché a pagare questo atteggiamento della maggioranza… *(Il

La Presidenza dichiara inammissibili gli emendamenti 5.0.2 e 8.5, ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento, in quanto privi di portata modificativa.

la stretta su chi guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di stupefacenti. Il punto è che andate ben oltre quella che è la limitazione a queste condizioni, poiché andate a rivedere un principio costituzionalmente garantito, che è quello della possibilità per il soggetto di dar prova di non essere in condizioni di non poter guidare, lo fate in maniera molto chiara andando a modificare l'articolo. L'emendamento soppressivo vuole ripristinare la condizione previgente dell'articolo in essere. Passando al merito,

possono dare dei risultati positivi ai *test* che vengono somministrati agli utenti della strada. Il soggetto che

Questo è un fatto noto sia ai medici sia ai giuristi che abbiamo ascoltato e che abbiamo voluto interpretare con questo emendamento soppressivo parziale. Inoltre, signor Presidente, vorrei ricordare che ho sottoscritto anche un emendamento del Gruppo AVS che va sempre in questo senso, per tutelare coloro che utilizzano dei medicinali ad uso esclusivamente terapeutico. Riteniamo ingiustificata la condanna e

parere è favorevole previa riformulazione dell'impegno come segue: tenuto conto prioritariamente delle esigenze di sicurezza della circolazione che impongono la previa verifica della idoneità psicofisica degli stessi».

«in condizione di disabilità»; quanto al terzo considerato, sostituire la parola «invalido» con le seguenti: «persona in condizioni di disabilità»; quanto all'impegno, sostituire con il seguente: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito delle modifiche al regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al DPR 16 dicembre 1992, n. 495, che, qualora la certificazione medico-legale dell'Azienda sanitaria locale di appartenenza attesti che le condizioni che danno luogo al rilascio dell'autorizzazione hanno carattere permanente o ingravescente e rientrano in una delle voci individuate dal decreto ministeriale 2 agosto 2007, tale autorizzazione ha carattere illimitato; di valutare, altresì, l'estensione della validità dell'autorizzazione a dieci anni, prevedendo l'introduzione di un codice QR e altre eventuali caratteristiche digitali che utilizzano mezzi elettronici con finalità antifrode».

Le Città 30 sono una visione di nuova mobilità sostenibile, già posta in essere in numerosi Comuni d'Italia

spingere sul pedale dell'acceleratore quando siamo in auto e corriamo per fare qualunque cosa. Città 30 è una visione che deve essere portata avanti e non deve essere smantellata, come invece il ministro Salvini sta facendo in quest'ultimo periodo. Più avanti magari interverrò nuovamente

nel momento in cui deve essergli sospesa la patente. I dati Istat rilevano che i soggetti che hanno meno di 20 punti sulla patente sono, allo stato attuale, pari a circa il 3 per cento della popolazione.

e tutti siamo convinti che il vero problema sia quello della sicurezza nelle strade - che il vero obiettivo del codice della strada debba essere quello di ridurre il numero degli incidenti e la mortalità, noi crediamo che il tema della formazione sia fondamentale.

ma davvero non volete cercare di incentivare il fattore culturale? Davvero possiamo pensare che, aumentando le pene, si risolvano i problemi della sicurezza stradale, senza cambiare la cultura con cui andiamo nelle strade, per la quale i nostri giovani sono abituati, fin da piccoli, a vedere le strade come qualcosa di altro da loro? *(Applausi)*. Vi chiediamo, dunque, di aumentate i corsi di formazione nelle scuole. Facciamola diventare una materia extracurricolare vera, facciamo approfondimenti e creiamo meccanismi per creare una nuova cultura sulla strada.

Scorrendo le pagine *social* del ministro Salvini posso affermare con sicurezza che questo articolo nasce proprio da quell'evento. Inizialmente il testo dell'articolo

di estendere da uno a tre anni l'attesa per un neopatentato di potersi mettere alla guida di un'auto

da uno a tre anni della limitazione nell'utilizzo delle auto più potenti da parte dei neopatentati,

potente. Tuttavia, sebbene quel testo avrebbe avuto un nostro voto favorevole, dopo questa inconcepibile modifica dichiaro il voto contrario del Gruppo MoVimento 5 Stelle.

agli aspiranti nuovi utenti della strada, coloro che conseguiranno la patente di guida, la possibilità di effettuare dei corsi

in quanto l'utenza deve essere messa nelle condizioni di sapere quali sono i fattori che possono generare minore sicurezza sulla strada, affinché possano essere affrontati e superati. Per questo dichiaro il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle.

e quando invece vengono assorbite. In questo caso, ad esempio, abbiamo votato l'emendamento 10.0.3, però lei non ha specificato che sarebbe stato votato insieme al 10.0.4; questo potrebbe trarre in confusione poi l'indicazione di voto che

semplicemente un ulteriore balzello per quelle società, ma probabilmente con quei numeri riuscirebbero tranquillamente a sostenerlo. Quello che ucciderà lo *sharing* sarà l'obbligo del casco per tutti, per tutti, anche per coloro che hanno acquisito grande dimestichezza nell'uso dei monopattini su strada. Lo dico perché a distanza di cinque anni, da quando si è sviluppato il grande mito del monopattino elettrico, diverse persone hanno iniziato ad utilizzarlo sin dai primi tempi. La

non uso il monopattino sui sampietrini, perché mi crea un problema alle braccia, mentre lo uso sulle strade lisce e asfaltate.

La persona che non ha voglia di pedalare, la persona che perde il bus o il cui autobus è perennemente in ritardo, sceglie di muoversi in maniera autonoma; la persona che non voleva pagare l'assicurazione del motorino, sceglieva di muoversi in monopattino.

Grazie a tutti motivi dei nostri emendamenti che voi avete appena respinto, ma questo mi serve solo per annunciare il voto contrario e giustificato del MoVimento 5 Stelle sull'articolo

l'articolo che ci stiamo apprestando a votare. Come senatrice con un lungo corso nell'ambito dell'amministrazione di Roma Capitale, so quante e quali sono state le difficoltà che abbiamo dovuto vivere con il precedente codice della strada. E rammento che, con l'attuale onorevole Matone, che era consigliere comunale insieme a me e insieme al relatore Andrea De Priamo, molte volte ci siamo dovuti misurare con il tema del decoro urbano relativo ai monopattini, alla mobilità dolce, al pericolo arrecato ai nostri giovani. Ricordo, per esempio, quante persone purtroppo hanno perso la vita per il fatto di andare in giro con Grazie a tutti

chiarezza - come sarebbe stato auspicabile e giusto - al tema della sicurezza dei cicloamatori e dei ciclisti sulle strade.

intenzione di rispettare le condizioni di sicurezza dell'utente più fragile.

bici). Un soggetto in auto è obbligato a rispettare il limite di un metro e mezzo nel sorpasso di una bici, perché è chiaro che l'autovettura crea uno spostamento d'aria e un risucchio che possono essere fatali per il ciclista. Le parole «ove le condizioni della strada lo consentano» vanno completamente a svilire l'intento della normativa. Sottosegretario, lo dico a lei perché, avendo seguito il provvedimento, avrà sviluppato anche lei una sensibilità

le associazioni che vi hanno chiesto di essere audite. Parlo di associazioni che rappresentano le vittime della strada, familiari e persone che hanno sofferto a causa di un incidente o una collisione del proprio familiare in bici con un'autovettura. I concetti erano ben chiari e

non andate ad aumentare la sicurezza sulla strada. State facendo finta di farlo, come avete fatto finta di ricevere le associazioni che vi chiedevano di essere ascoltate per ottenere davvero una maggiore sicurezza sulla strada. I dati ce lo confermano; non stiamo andando in questa direzione. Ci sono Ci sono situazioni simili, applicate già in altri Paesi europei, che riportano statisticamente il miglioramento delle incidentalità sulla strada. C'è il Piano nazionale sicurezza stradale, di derivazione europea, che ci invita a tendere, entro il 2030, a zero morti in Il ministro Salvini ha detto che sta andando in questa direzione anche con questo provvedimento, ma a noi non risulta. Continueremo a intervenire anche per dare voce alle persone che fuori da queste Aule ci stanno contattando e stanno manifestando. Sono giorni che riceviamo *e-mail*:

veicoli destinati al trasporto di persone e merci già circolanti, che ad oggi non sono soggetti all'obbligo dell'installazione di dispositivi

di avvicinamento di un soggetto vulnerabile, che non si rende conto della sagoma di questi mezzi così voluminosi. In Commissione questo emendamento è stato trasformato in ordine del giorno ed è stato accolto dal Governo. Io volevo approfittare

per far sì che questo ordine del giorno diventi realtà, è necessario istituire un fondo affinché i soggetti proprietari possano essere aiutati, almeno in parte, nell'installazione di questi nuovi dispositivi. È certamente un'innovazione legislativa che va a migliorare, questa

Presidente, e vorrei evidenziare all'Assemblea l'importanza di un voto favorevole su questo ordine del giorno. Stiamo parlando della realizzazione dei corridoi faunistici. Sul nostro territorio, le poche aree verdi e naturali che sono rimaste - e che sono tutelate - sono spesso attraversate da infrastrutture stradali. Questo sicuramente rende piacevole il viaggio, guardando a destra e a sinistra prati e boschi, ma non si considera che in quei prati e in quei boschi vivono animali, ossia la fauna selvatica. La presenza dell'infrastruttura crea un ostacolo agli spostamenti della fauna selvatica. Esistono dei corridori naturali (sono cunicoli che passano sotto queste strade), che però, a causa anche degli eventi atmosferici, si occludono;

abbiamo deciso di partecipare a un progetto europeo di ripopolazione dell'orso bruno. Tra le condizioni previste dal progetto vi era la creazione dei corridoi faunistici, proprio immaginando che questi orsi si sarebbero spostati nelle aree più interne per ricongiungersi con altre popolazioni di orsi già presenti. Purtroppo questo progetto è stato accettato, è stato sottoscritto, sono stati

si impegna il Governo, laddove ci fossero dei fondi disponibili, a destinarli alle risorse necessarie per realizzare una rotatoria in corrispondenza dell'incrocio tra via Basse del Brenta e via Michela, stazione, strada provinciale 24. Io sono andato a vedere su Google Map: effettivamente c'è lo spazio per costruire una rotatoria, perché accanto c'è una fattoria però mi sembra che anche più avanti ci siano altri posti che si prestano alla rotatoria. Allora facciamo un elenco di ordini del giorno su Google Map e ciascuno di noi può dare dei suggerimenti su dove fare delle rotatorie, che mi sembra anche pertinente a quello di cui stiamo discutendo.

Signora Presidente, intervengo per sottolineare il senso di questi emendamenti soppressivi che il Gruppo ha presentato. pensiamo che questa sia una grande occasione persa. Lo dico perché questa raffica di votazioni, signora Presidente, rischia di farci perdere il senso profondo di questa riforma del codice della strada. Doveva essere l'occasione

che i maggiori pericoli per i pedoni, per i nostri figli e per i nostri anziani si trovano proprio nei tessuti urbani. Questa era una grandissima occasione. Quando l'associazione dei familiari delle vittime della strada dice

bene prima, così come è stata sottolineata la limitazione alla scelta della mobilità sostenibile. Ma io vorrei intervenire, signora Presidente, per sottolineare un altro aspetto, in particolare agli amici della Lega.

mentre il Presidente degli Stati Uniti neoeletto pensa a mettere i dazi contro l'Europa, noi stiamo pensando di delegare il commercio estero al Veneto. Questo è il senso dell'autonomia.

non ha né capo né coda, impostato così. Bisognava dare più autonomia ai sindaci, non meno autonomia, non più libertà a ognuno di fare quel che gli pare nel tessuto urbano, togliendo le sanzioni multiple. Bisognava responsabilizzare gli utenti. E chi la fa chi la fa quest'opera? Un funzionario del Ministero delle infrastrutture? Ma via, ma siamo seri, dai. Questo provvedimento, impostato così, è

senza avere la possibilità di fare alcuna modifica. Ora ci stiamo accingendo a votare l'articolo 35, che è una delega per modificare tutto quello che fino a qui abbiamo discusso e votato. Una delega che, a detta del collega Rosso, che ieri, in discussione generale, ci ha raccontato quello che sarà il nuovo codice della strada, darà un testo completamente diverso da tutti i 34 articoli che abbiamo fino adesso discusso e votato.

come prevede la normativa europea, inserire la tecnologia per controllare gli angoli ciechi dei TIR e dei grandi e dei grandi veicoli, che sono la principale fonte di incidenti, anche mortali. Stiamo chiedendo di utilizzare una tecnologia

la possibilità di inserire la tecnologia, la formazione. Altrimenti, questo nuovo codice della strada, non solo non porterà a nulla, ma sarà foriero di tanti incidenti e, purtroppo, di tante nuove morti.

Ricordiamo, però, che qui stiamo parlando di persone con una disabilità permanente, alle quali viene richiesta, nonostante la certificazione INPS, di rinnovare ogni cinque anni tale certificazione, per per verificare se possono avere delle agevolazioni rispetto alla sosta o rispetto alla circolazione. Con questo ordine del giorno, noi chiediamo al Governo, se la disabilità è certificata ed è

Signora Presidente, mi ha colto in contropiede, non mi aspettavo questa solerzia, ma la ringrazio comunque. Presidente, ci accingiamo a votare un provvedimento che tocca la vita delle persone ed è chiaro che non uso questo termine a caso. A differenza di altri Paesi, infatti, in Italia permane ancora una sottovalutazione sociale diffusa sul mettersi alla guida dopo aver bevuto, sul mancato rispetto dei limiti di velocità in città, sull'uso dei cellulari. C'è un detto che ricorre tra gli utenti della strada: negli altri Paesi le regole del codice della strada sono regole, da noi sono consigli per l'uso. Non è così, purtroppo; dovrebbero essere regole anche da noi, ma nella testa delle persone questo non è ancora entrato. Cito non a caso i comportamenti di cui sopra, percepiti come peccati veniali e che invece sono tra le principali cause degli incidenti, anche mortali. Ieri la collega Zampa ricordava alcuni dati: gli incidenti stradali sono la principale causa di morte tra gli *under* 30; il tasso di mortalità stradale in Italia è due volte maggiore di quello del Regno Unito e molto più alto di quelli della Germania, della Spagna e della Francia. C'è poi il danno economico, che si salda alla tragedia sociale: quasi 18 miliardi di euro nel 2022, ovvero quasi un miliardo del PIL. Davanti a tutto questo, Presidente, noi ci aspettavamo un provvedimento che puntasse con decisione verso la prevenzione. prevenire non significa solo fare campagne di sensibilizzazione, che comunque sono importanti; significa anche garantire la manutenzione delle strade, favorire la mobilità alternativa, l'uso dei mezzi pubblici, la presenza dei taxi nelle ore notturne e quant'altro possa servire per consentire una mobilità più *soft* e meno a rischio. Significa ridurre la presenza e la circolazione di auto nelle nostre città e di ridurne la velocità. Significa anche avviare una riflessione sugli esami per il rilascio delle patenti, perché la sensazione è che troppo spesso si sia di manica generosa, e questo al netto delle truffe sui rilasci e sui rinnovi che ogni tanto leggiamo sui giornali. Questo testo, invece, è in scia con lo spirito che anima il Governo attuale di fronte di qualsiasi questione sociale. Si inaspriscono le pene, si aumentano le sanzioni, si cerca come sempre il nemico da additare, il capro espiatorio responsabile di ogni male: chi sbaglia è colpevole, ma non si va a scavare sul perché qualcuno sbagli, che è il vero problema. Certo che i comportamenti incivili e incoscienti vanno condannati e perseguiti, questo nessuno lo discute, ma non diminuisci gli incidenti se continui a immaginare una mobilità auto-centrica, se restringi le norme a tutela dei bambini, degli anziani e dei ciclisti, se rendi più difficile mettere in sicurezza i marciapiedi, le piste ciclabili, le zone a traffico limitato, se non investi in miglioramento delle infrastrutture. Il punto vero, Presidente, è che questo provvedimento sgancia brutalmente la sicurezza stradale dal tema più generale della transizione ecologica a questo riguardo nel provvedimento che abbiamo letto. È un provvedimento centralista, perché toglie potere ai sindaci, al loro lavoro per ripensare le città in una chiave di sostenibilità urbanistica e di tutela dei soggetti più fragili. Insomma, la sensazione alquanto amara è più dell'ennesima occasione mancata: è un provvedimento ideologico, come sempre debole con i forti e forte coi deboli, come l'hanno definito le associazioni dei familiari delle vittime della strada all'uopo audite.

di porre fine innanzitutto umanamente, o quantomeno di tentare di arginare con gli strumenti nei nostri poteri che sono le norme, al triste e quotidiano *countdown* di morti e incidenti sulle arterie stradali del nostro Paese. Un impegno che avevamo assunto nei confronti di tutti gli utenti della strada, soprattutto i vulnerabili, traguardo che la dice lunga sull'impegno con gli italiani del Governo Meloni e del ministro Salvini, dopo trent'anni dall'ultima riforma del codice della strada. Correva infatti l'anno 1992. Solo questo potrebbe bastare a darci la misura ed il senso di questa riforma organica tanto attesa, che siamo certi renderà le nostre strade più sicure e più moderne dopo anni di inerzia e di interventi spot, *alias* propagandistici, capaci di alimentare soltanto il caos sulle nostre strade. Al contrario, con questo nuovo codice della strada vogliamo ridare armonia ed equilibrio a norme per certi versi obsolete, non più attuali, adattandole alle esigenze che la realtà di oggi ci impone. Una realtà che vede le nostre strade maggiormente percorse e, come dicevo, purtroppo un aumento esponenziale di incidenti, spesso, troppo spesso, coinvolgono giovani e giovanissimi. Spiace davvero, Presidente, assistere al solito teatrino di chi continua a negare la bontà e la necessità di alcune misure non più rinviabili, se vogliamo davvero contrastare la lunga sequela di morti sulle nostre strade e garantire così una mobilità più sicura a tutti i cittadini, perché è proprio questo l'obiettivo del disegno di legge che stiamo per approvare: contrastare senza se e senza ma le principali cause di incidenti stradali, rendere le strade più sicure e assicurare alla giustizia, con pene che siano correttamente severe, chi commette o addirittura reitera reati stradali. In altri termini, non possono esistere, signora Presidente, vie di mezzo quando si parla di sicurezza stradale, ma deve esistere tolleranza zero - e ne siamo molto orgogliosi - contro chi, recidivo, continua a mettersi alla guida ubriaco o dopo aver assunto sostanze stupefacenti e serve stupefacenti e serve pugno duro, durissimo, contro chi usa il cellulare alla guida: una pessima abitudine che fatica ad abbandonarci ancora oggi e che rappresenta una delle principali distrazioni, ovvero la primissima causa dell'incidentalità. Vieni beccato con il cellulare alla guida? Ti ritiriamo e sospendiamo immediatamente la patente sin dalla prima infrazione, senza se e senza ma, come pure se passi con il semaforo rosso, o non dai la precedenza ai pedoni negli attraversamenti pedonali, ti verrà ritirata la patente da un massimo di sette anni ad un minimo di quindici giorni. minimo di quindici giorni. Questa è certezza di vera sicurezza stradale. Non solo, però, repressioni delle infrazioni più gravi. Ci teniamo, Presidente, anche a fare prevenzione, grazie a quei corsi di educazione stradale rivolti ai giovani e giovanissimi, per responsabilizzarli sui rischi e sui pericoli di certe condotte, perché quella che abbiamo intrapreso a favore della sicurezza stradale sia davvero una battaglia di civiltà e - lasciatemi pure dire - di educazione civica, soprattutto di educazione civica. Non possiamo infatti ignorare che, da quando la mattina usciamo di casa fino a quando vi rientriamo la sera, siamo tutti utenti delle nostre strade. Per questo motivo il nuovo codice della strada ci riguarda ci riguarda tutti. Basta leggere i dati diffusi dall'Istat e dalla Polizia di Stato per rendersene conto. Oggi le principali cause di incidente stradale sono la distrazione, il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata, mentre la guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione per l'uso di sostanze stupefacenti era e rimane uno dei comportamenti più pericolosi in assoluto. Per questo - come annunciavo prima e ci tengo a ribadirlo a chi ci sta ascoltando da casa - andiamo a contrastare questo odioso e irresponsabile fenomeno alla guida, un fenomeno tristemente capace di lasciare una lunghissima scia di sangue dietro di sé. Un fenomeno che ci deve coinvolgere tutti, come persone prima che come legislatori, perché ancora troppe famiglie piangono i propri figli, uccisi da chi poteva e soprattutto doveva evitare di mettersi alla guida di un'automobile, divenuta a quel punto strumento inesorabile di morte, con un telefonino. I recidivi, cioè coloro che sono già stati condannati per aver guidato con un tasso alcolemico superiore ai limiti imposti per legge, si vedranno comminare il divieto assoluto di assumere bevande alcoliche e, nei casi più gravi di recidiva, si potrà guidare solo dopo aver installato sul veicolo, a spese dell'interessato, l'*alcolock*, un dispositivo che impedisce al mezzo di avviarsi qualora venga riscontrato un tasso alcolemico del guidatore anche di poco superiore allo zero. Questo significa avere un pugno duro, sì, perché la vita è il valore più grande che il Governo è chiamato a tutelare e ne siamo orgogliosi. Questa per noi - lo ribadisco - è la differenza tra battersi il pugno sul petto per la disperazione e garantire viceversa la sicurezza stradale. Sono poi commossa e ringrazio il ministro Salvini per la sensibilità dimostrata nell'aver fatto propria una norma della quale avevamo discusso nel corso del mio *question time* sulla gestione degli animali domestici. Voglio dire un grazie sentito alla senatrice De Girolamo, per aver sottoscritto questo articolo,

che ci sia un altro atteggiamento da parte di chi è chiamato a fare delle delibere a favore degli animali domestici in questo Parlamento, perché ci si mette semplicemente sentire* con il sentimento della gente e soprattutto con il sentimento in questo caso dell'Assemblea. Il ritiro della patente e l'inasprimento delle pene contro chi abbandona gli animali in strada è per me una norma sovrana; un reato, prima ancora che un fenomeno, altrettanto odioso, vigliacco, bieco e feroce, perché commesso su esseri indifesi e - attenzione - su esseri senzienti, che provano sentimenti e dolori. Quindi è giusto che non vengano trattati come oggetti, come fanno quegli orrendi criminali che abbandonano i nostri animali per strada, abbandonandoli al loro destino, abbandonandoli alla sofferenza e spesso causando Grazie a tutti gettati sui marciapiedi e sulle piste ciclabili, a intralciare pedoni e mezzi di soccorso, sporchi, incidentati, distrutti. Ora chi li utilizza dovrà rispettare il codice della strada, invece, e dotarsi di contrassegno di assicurazione; non potrà uscire dai centri abitati e obbligatoriamente dovrà indossare un casco. Nessun furore ideologico, colleghi; servivano semplicemente Grazie a tutti

dalle associazioni di categoria, e anche a quella norma che dico essere di civiltà sugli autovelox o i T-Red di nuova installazione, grazie a cui avere il conto alla rovescia e una durata minima del giallo, perché tali strumenti non siano dei semplici bancomat a danno dei cittadini e a solo vantaggio dei Comuni che vogliono fare cassa. Da ultimo, abbiamo voluto riportare ordine su delle norme in certi casi dettate da certi sindaci semplicemente per propaganda e furore ideologico, questo sì (e chiudo quasi, Presidente). Mi riferisco alle cosiddette Zone 30 del nuovo codice. Vogliamo allora dire un sì forte e convinto alle Zone 30 vicine ad asili, scuole, campi sportivi, ospedali, parchi giochi; un altro forte sì alle Zone 30 nelle strade senza marciapiedi o dove c'è intenso traffico di pedoni e ciclisti. un secco no, invece, a tutte quelle ordinanze illogiche, prima ancora che ideologiche, che vorrebbero imporre i 30 chilometri orari nelle nostre città, tradendo lo spirito della norma e mettendo in difficoltà i cittadini senza il minimo beneficio in termini di sicurezza e di riduzione delle emissioni, e probabilmente anche le aziende produttrici, perché sono norme che sottendono all'idea di eliminare i parchi veicoli dalle nostre strade. Concludo allora, signor Presidente, dicendo che la sicurezza e la tutela dell'ambiente e della salute delle persone fragili, coniugate con la modernità, l'efficienza, la sostenibilità e il buonsenso, fanno da cardine a questa riforma indispensabile per la quotidianità degli italiani. Siamo orgogliosi di poter andare avanti in questa direzione, al fianco del Governo Meloni, nel combattere questa epocale battaglia in nome della vita e della sicurezza stradale, per la sicurezza dei nostri figli e per la sicurezza di tutti noi utenti della strada. Questo è il sentimento che ci ha accompagnato nel costruire un provvedimento non più rinviabile e che voteremo convintamente. Ogni morto in meno, ogni candela in meno, ogni fiore in meno sulle nostre strade darà un senso superiore al nostro essere qui in queste solenni Aule non ad occupare semplicemente degli scranni, ma a garantire il futuro dei cittadini.

non vediamo una definizione complessiva di che cosa si vuole fare effettivamente per la sicurezza. Ci sono alcune norme

uscendo da una discoteca prenda un'auto e succeda l'irrimediabile, come ogni sabato sera purtroppo ci dicono le cronache delle nostre città che si riempiono di morti. Ad esempio, banalmente

la quale sono sottodimensionati e non riescono a fare i controlli. Analogamente, si parla di controllo della velocità ma poi si depotenzia l'utilizzo degli autovelox, perché vengono considerati strumenti per fare cassa. Allora delle due l'una: o mettiamo gli autovelox o mettiamo la Polizia stradale. Come si fa a controllare una persona che ha assunto delle sostanze stupefacenti o alcoliche che si mette alla guida di un'autovettura? Non c'è una cornice ideale in questo codice della strada per evitare i morti. Evidentemente se ne sono accorti anche i soggetti che da anni si occupano di questo argomento: ventisei associazioni di familiari di familiari di vittime della strada hanno scritto ripetutamente in questi giorni a noi senatori per dire di porre rimedio a questo codice che non ha avuto una lettura seria al Senato, perché non sono state apportate rilevanti modifiche rispetto a quello che era accaduto alla Camera. Eppure, essendo un codice e non un decreto che decade, si sarebbe potuto incidere molto di più dopo aver ricevuto delle sollecitazioni da parte di chi per anni si è occupato di tutelare la memoria delle proprie vittime, ma soprattutto facendo atti concreti contro quella che viene definita una mattanza quotidiana. Siamo ormai arrivati a oltre 3.000 morti sulle strade e più di 250.000 feriti, soltanto quest'anno: è veramente una tragedia infinita che non vede riscontri in norme adeguate. Viene veramente da sorridere perché questo Governo, che difendeva con la sua maggioranza la bontà dell'autonomia differenziata non più tardi di ieri (non è che stiamo parlando di interventi fatti a inizio legislatura), e che anzi di fatto dice come la Corte costituzionale abbia mantenuto integra l'autonomia differenziata e quanto sia importante dare voce alle Regioni e agli enti locali, stabilisce centralmente quali possono essere le Zone a traffico limitato e le Zone 30. Ma un sindaco non è in grado di stabilire nella sua città quali sono i luoghi dove mettere le ZTL e le Zone 30? Inoltre, se i cittadini non saranno contenti delle scelte che, come diceva prima la collega, sono dettate da furore ideologico, banalmente, cinque anni dopo Non credo che un sindaco abbia bisogno di un tutore romano che non conosce la città e che non sa quali sono gli elementi necessari per dare una svolta ecologica anche alla città, perché le Zone 30 servono anche a diminuire le emissioni in atmosfera. Nel provvedimento non c'è nulla per un'alternativa vera all'autovettura, perché, al netto della sicurezza data ai monopattini, invece molto poco viene fatto per incrementare le piste ciclabili e la possibilità di andare avanti per quanto riguarda…

eletto dai cittadini; poi ripeto che, se i cittadini non saranno contenti delle scelte fatte a livello comunale per stabilire quali sono le ZTL e quali sono le Zone 30, manderanno a casa felici e contenti questo sindaco incapace e pieno di furore ideologico, altrimenti banalmente verrà riconfermato. Visto che, quando ci fu il furore ideologico, era stato

non soltanto di mezzi pubblici, ma già di mezzi privati: ci sono le autovetture che si possono guidare da minorenni, i motocicli, le biciclette e i monopattini. Non sono solo soggetti che vengono scarrozzati, ma sono loro stesse persone che guidano e devono essere in grado di capire che utilizzare un cellulare mentre si guida non va bene,

tipiche, ahimè, del Ministro che ha partorito questo codice della strada, cioè il ministro Salvini, che ha inasprito un po' le pene, ha inasprito un po' le multe, ma poi di fatto ha annacquato la possibilità di fare la differenza nel codice, perché tendenzialmente sarebbe andato contro a quelli che lui probabilmente pensa essere i suoi elettori ideali, cioè quelli che vogliono meno regole, meno lacciuoli, per poter essere liberi e perché devono fare un po' quello che desiderano. Per questo motivi e per dare voce alle lettere che in questi giorni abbiamo ricevuto perché venissero posti in essere degli emendamenti, non perché venisse del tutto stracciato questo ma perché venissero ascoltati veramente i soggetti che in questi anni, sulla loro pelle, hanno vissuto delle tragedie, noi abbiamo orgogliosamente votato contro ogni articolo, perché non avevano

purtroppo nel 2023 sono ancora 3.039 i morti in incidenti stradali in Italia. Che otto persone al giorno muoiano ancora sulla strada, nonostante i passi avanti che sono stati fatti in tema di sicurezza, è preoccupante e merita nuove norme restrittive. Le vittime aumentano anche per i conducenti di monopattini (sono state 21 nel 2023) e per le biciclette (sono state 212). Il confronto con l'Unione europea è impietoso: per ogni milione di abitanti si contano in media 45 morti nell'Unione europea, mentre nel nostro Paese sono ben 52. Rimaniamo purtroppo al diciannovesimo posto in Europa. Infine, su più di 52.000 incidenti con lesioni sono 5.085 quelli con almeno un conducente in stato di ebbrezza e 1.700 quelli con un conducente sotto effetto di stupefacenti. E per le sanzioni rimangono ai primi posti l'eccesso di velocità e l'utilizzo durante la guida di *smartphone*. Nel complesso, sono dati molto preoccupanti. Questo disegno di legge dà risposte proprio a questi problemi, inasprendo le norme e le sanzioni, anche penali, sulla guida in stato di alterazione psicofisica, sull'omicidio stradale, le lesioni stradali, i superamenti dei limiti di velocità: una stretta assolutamente necessaria per salvare vite. Così come viene rivisitato il sistema della patente a punti, dopo una decurtazione che porti il titolare ad avere meno di 20 punti, oltre all'ulteriore decurtazione del punteggio residuo viene irrogata anche la sanzione della sospensione breve della patente. Ma investiamo anche nella prevenzione, attraverso la formazione dei guidatori, così come inseriamo una maggiore gradualità alla guida delle cilindrate maggiori per i neopatentati. Grande attenzione è stata dedicata ad aumentare la sicurezza delle biciclette e dei veicoli di micromobilità elettrica. Alle modifiche che introducemmo nel 2021 in Commissione trasporti alla Camera (segnalatori di direzione, freni, velocità massima a 20 all'ora, giubbotto catarifrangente di notte), si aggiungono ora casco, assicurazione e targa. Vista la complessità della materia, il disegno di legge comprende un'ampia delega legislativa per il riordino complessivo della materia stessa. Sono stati numerosi gli emendamenti di Forza Italia approvati alla Camera, e anche qui al Senato abbiamo presentato un pacchetto importante di emendamenti volto a migliorare ulteriormente il testo nella direzione della sicurezza e della prevenzione. In considerazione dell'urgenza di entrare in vigore che hanno molte disposizioni salvavita contenute in questo disegno di legge, abbiamo convenuto che un nuovo passaggio alla Camera ne avrebbe rinviato troppo l'entrata in vigore, per questo motivo abbiamo ritenuto di convertire gli emendamenti più significativi in ordini del giorno che impegnano il Governo a inserirne il contenuto e il dispositivo nei decreti di attuazione della delega. Abbiamo quindi impegnato il Governo, con questa serie di ordini del giorno, a rivedere la disciplina speciale relativa ai neopatentati e a dare attuazione all'insegnamento a scuola guida degli effetti di alcol e droga sulla guida, di elementi di primo soccorso, dei fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada. Abbiamo impegnato il Governo a rivedere la materia della destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni irrogate per le violazioni al codice della strada, assicurando la destinazione prioritaria alla sicurezza stradale, alla manutenzione delle strade, all'aggiornamento della segnaletica e non solo per tappare buchi di bilancio. Si dovranno adottare misure per l'installazione dei dispositivi di segnalazione della sagoma dei mezzi pesanti adibiti a trasporto collettivo di persone, cioè dei pullman. Lo abbiamo già fatto con i TIR e l'Europa ci ha copiati; ora ora chiediamo che venga fatto anche per i pullman. L'articolo 35 collega la dissuasività della sanzione anche alle situazioni reddituali del soggetto. Abbiamo voluto specificare che, in sede di attuazione della delega, questo principio venga interpretato non nel senso di alzare le sanzioni a chi ha un reddito più elevato, mantenendole immutate per i meno abbienti, ma invece di ridurre l'importo delle sanzioni per i meno abbienti, mantenendo le altre immutate. Si dovranno promuovere meccanismi di avviso digitale finalizzati a segnalare la scadenza della patente di guida, con modalità semplificate per l'utente; prevedere un importo massimo per tutta Italia da corrispondere per l'accesso alle ZTL. Abbiamo impegnato il Governo ad adottare disposizioni volte a individuare una soglia della sanzione pecuniaria al di sotto della quale non è dovuto il versamento del contributo unificato e comunque prevedere la restituzione dello stesso in caso di accoglimento accoglimento dell'opposizione. Abbiamo proposto di individuare meccanismi premiali che incentivino il trasgressore al pagamento della sanzione in tempi estremamente ridotti, anche prevedendo una riduzione più alta dell'importo della sanzione prevista. Per quanto riguarda la micromobilità, abbiamo lavorato per rendere le nuove norme più eque. Siamo intervenuti per far sì che l'assicurazione dei monopattini sia di costo adeguato alla lesività del mezzo, sicuramente inferiore ai veicoli di maggiore potenza come le auto o i camion. sul casco obbligatorio per i monopattini ci siamo chiesti come mai non fosse stato introdotto anche per le biciclette, stante i dati di mortalità 212 deceduti per le biciclette e 21 per i monopattini. Ricordo che attualmente è ancora consentito a un minore di condurre una bicicletta di notte su una strada extraurbana senza un casco protettivo. Il casco obbligatorio anche per i minorenni anche per i minorenni potrebbe indurre anche gli adulti ad adeguarsi, come è successo, per esempio, per il casco obbligatorio per i minori sulle piste da sci. Pensate che su 50 bambini deceduti nel 2023, 6 erano in bicicletta. Anche su questo argomento il Governo ci ha ascoltato e si è impegnato in sede di delega a perseguire l'obiettivo della sicurezza della circolazione, con particolare riguardo all'uso di sistemi di protezione personale da valutare in relazione alle caratteristiche tecniche e all'utilizzo dei velocipedi. Abbiamo infine fatto presente le difficoltà delle aziende di *sharing* ad adeguarsi alla normativa del casco, ricordando che ci sono oltre 5.000 lavoratori a rischio. Anche in questo caso il Governo si è impegnato a valutare l'impatto della misura. Siamo soddisfatti sia del fatto che anche il Senato abbia potuto approfondire tematiche che interessano la vita quotidiana di tutti gli italiani, sia che il Governo abbia riconosciuto la validità delle nostre proposte e osservazioni. Voglio essere chiaro perché ho ascoltato tutto il dibattito di ieri: oggi voteremo convintamente questo provvedimento. Le proposte fatte da Forza Italia non toccano le norme che entreranno subito in vigore, ma vedranno la luce in fase di delega, non stravolgendo, ma rafforzando il provvedimento. Sono convinto che abbiamo lavorato duramente per migliorare la sicurezza di tutti e per ridurre quei lutti improvvisi e strazianti che ancora troppe famiglie provano tutti i giorni.

ieri in discussione generale ho voluto dare voce alle associazioni delle vittime sulle strade che di fatto - voglio essere anche oggi chiara e netta hanno subito la tremenda e disumana strumentalizzazione da parte del ministro Salvini e della maggioranza in merito al provvedimento sul codice della strada. Il ministro Salvini ha avuto il coraggio di legare il nuovo codice della strada ad una sorta di omaggio alle vittime di incidenti stradali e alle loro famiglie. Ieri pomeriggio, anche in quest'Aula, ho dovuto sentire esternazioni veramente imbarazzanti e fuori luogo. La destra afferma che questo codice della strada salverà vite umane. Viviamo sullo stesso pianeta?

Dopo quello che è stato detto ieri da alcuni esponenti della destra come Potenti e Pellegrini, potremmo quasi dire che parte della maggioranza in quest'Aula è stata un'incubatrice di *fake news*. Le associazioni delle vittime sulla strada si sono dovute scomodare per dichiarare pubblicamente che lo sfregio ai familiari delle vittime di violenza stradale è doppio e inaccettabile. Ieri avete avuto il coraggio di cavalcare il dolore di chi oggi non ha più voce, perché vittima di un incidente stradale, e lo state facendo anche oggi. Avete cavalcato anche la sofferenza di intere famiglie straziate da lutti dovuti a questi incidenti, famiglie che in un istante hanno perso persone amate, amiche, giovani e meno giovani, bambine e bambini. Sappiamo con certezza che nessuna raccomandazione o richiesta presentata dalle associazioni dei familiari delle vittime è stata accolta. Zero. È francamente inaccettabile sentire anche in quest'Aula, anche oggi, quanto poco vi interessi la realtà dei fatti, evidentemente per il vostro tornaconto elettorale. C'è un motivo per cui il codice della strada è stato soprannominato codice della strage. O credete veramente che le associazioni delle vittime si siano svegliate una mattina, decidendo di chiamarlo così, a caso, per sfizio, per gioco, per divertimento? Che opinione avete del lavoro che quotidianamente fanno per educare e formare alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile? Tutte le associazioni delle vittime sulla strada, centinaia di persone esperte del settore, si sono pronunciate contro questo codice e a microfoni e telecamere spente persino la maggioranza si permette di dire che alcuni articoli sono inaccettabili. Eppure ciò non si rispecchia nel vostro voto. voto. Anche oggi, a maggior ragione in presenza del ministro Salvini, ritengo importante dare di nuovo voce direttamente a Marco Scarponi della Fondazione Michele Scarponi, familiare di una vittima della strada, famoso ciclista su strada che vinse anche il Giro d'Italia nel 2011 e che è morto in un incidente stradale, investito da un furgone mentre si stava allenando sulle sue strade che conosceva come le proprie tasche. Parlo di una delle associazioni che il ministro Salvini si è più volte vantato di aver ascoltato. Rileggo, anche per le colleghe e i colleghi che ieri non hanno potuto partecipare alla discussione generale, Marco Scarponi: «Onorevole Ministro, tanti familiari delle vittime, come me, i miei genitori e mia sorella, non hanno scelto di diventare quello che sono oggi. La tragedia che ci ha colpito sette anni fa con la morte di Michele ci ha portato a reagire impegnandoci ogni giorno per una nuova strada che salvaguardi più vite umane possibili. Noi e tanti come noi abbiamo creato associazioni e fondazioni, entriamo nelle scuole, promuoviamo occasioni di confronto e incontriamo cittadini e cittadine ogni giorno. Alcuni di noi sono diventati veri e propri tecnici della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile. Se qualcosa è cambiato in meglio in merito a questi aspetti nel nostro Paese, lo dobbiamo anche a loro. Abbiamo aspettato tanto tempo, troppo, che il codice della strada, quel patto stretto tra tutti noi per condividere la strada in pace, cambiasse, mettendo al centro finalmente una visione giusta, nuova, con la persona e la vita al primo posto e con tutte quelle riforme necessarie per favorire una vera cultura della della sicurezza stradale e della mobilità attiva e sostenibile. Confidavamo davvero che queste modifiche fossero una risposta a un passato e a un presente ancora di dolore e ci aprissero un futuro di speranza. Purtroppo non è così. Non è corretto che il Governo dica che ha ascoltato le associazioni dei familiari delle vittime. Le ha fatte parlare, ma non le ha ascoltate, non ha preso niente di quanto è stato detto nelle audizioni. Questo atteggiamento non solo tradisce le aspettative di chi crede in una mobilità più sicura, ma ferisce profondamente coloro che hanno già pagato un prezzo altissimo. Marco Scarponi». Le associazioni sono state barbaramente strumentalizzate. Questo è. Colleghe e colleghi della maggioranza, quando voterete questo codice della strada dovrete essere perfettamente consapevoli che voterete contro le associazioni dei familiari delle vittime sulla strada, ma anche contro le future generazioni, tra cui anche le nostre figlie e i nostri figli che tanto volete punire per le loro scorrette azioni, anche con questo codice della strada, e che hanno invece il diritto di circolare in sicurezza tutti i giorni sulle nostre strade che anche voi sapete essere spesso molto pericolose. In più ieri, in discussione generale, siamo venuti a conoscere altri nemici che ha la destra. Per la destra ci sono vecchi e nuovi nemici ad ogni angolo: prima gli immigrati, poi gli ambientalisti e ancora le donne e i loro diritti. Adesso i nemici sono i giovani: bravi e belli quando lavorano sottopagati e si accontentano di otto metri quadri di stanza a 1.000 euro di affitto al mese; terribili e da incarcerare quando chiedono più diritti per le persone e per il pianeta. Ieri il senatore Potenti ha dato dei gradassi e degli irresponsabili ai giovani; la senatrice Pellegrino ha parlato di ragazzi drogati, ubriachi, in stato di ebbrezza, che pensano solo allo sballo. Ma cosa vi hanno fatto di male questi giovani? Perché continuate a denigrarli e a colpirli nei diversi provvedimenti che portate in Aula, dal disegno di legge sicurezza al decreto rave, solo per citarne due? Dai vostri interventi di ieri sembra che siano proprio loro i principali responsabili degli incidenti in Italia e che per questo servano misure repressive forti con i deboli e deboli con i forti. Ieri ho voluto controllare i dati. Secondo i dati ACI-Istat del 2023, la fascia d'età dei giovani è responsabile di circa il 10-12 per cento degli incidenti stradali con lesioni a persone in Italia. Che si fa con il restante 88 per cento? Veramente volete continuare a criminalizzare un'intera fascia di popolazione? Perché non entrate o non siete entrati anche in qui in Aula nel merito del vero problema della sicurezza sulla strada,

avete preferito dare tutta una serie di diritti pericolosi proprio ai veicoli a motore. Avete deciso di allentare alcune restrizioni e dare loro maggiore libertà di circolare, permettendo maggiore velocità anche alle giovani generazioni, che poi però andrete a castigare, e riducendo controlli e sanzioni. Ieri, in Ieri, in discussione generale, avete illustrato molto bene la visione antiquata che avete della circolazione, della sicurezza futura delle strade italiane e della mobilità sostenibile. Oggi, voi della maggioranza, con questo codice della strada votate il ritorno a un passato pericoloso, un via libera alla giungla urbana, una minaccia per tutte e tutti: automobilisti, pedoni, ciclisti, famiglie, persone con disabilità e comunità intere. Per quanto riguarda il lavoro in Commissione, non so come qualcuno possa aver affermato che abbiamo lavorato in sintonia, quando non c'è stato alcun margine di azione per migliorare il testo, ma solo finta e mielosa apertura al dialogo. Sembrava che alcuni emendamenti si sarebbero potuti trasformare in ordini del giorno che sono stati stati poi definiti non vincolanti. Peccato, però, che il *Diktat* del Governo sia stato di non toccare i punti cardine del disegno di legge, proprio quelli più problematici sulla sicurezza e l'incolumità della strada. Io spero ancora che oggi siate in grado di immedesimarvi in una studentessa che va all'università o a scuola in bicicletta con il terrore di essere schiacciata da un camion e dai suoi angoli ciechi. Spero possiate immedesimarvi, per un solo momento, in una persona che perde un proprio caro: provate a immaginarlo solo un istante e non voterete questo codice della strada. Noi non possiamo rassegnarci. La vita non è uno scherzo e va presa sul serio. Non vogliamo continuare a guardare dalla finestra, senza far niente, quelle città europee e qualche città italiana virtuosa, come Bologna, che invece stanno creando spazio per grandi e piccoli, per i cittadini, facendo tornare a vivere strade e piazze, facendo crescere la qualità di vita nonché l'economia locale, restituendo la città alle persone.

con un *iter* procedurale molto snello, affinché entro agosto si avesse il nuovo codice della strada revisionato. Così però non è stato, perché, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, c'è stato uno *stop*. Questo probabilmente perché

Allora, Ministro, sa cosa le dico? Le parole contano tanto e contano molto di più di quelle che vengono usate negli *spot* o nei *post*. Questo lo dico anche in ragione del fatto che i dati di rilevamento del tasso degli incidenti stradali riguardano davvero tutti i cittadini e tutti i santi giorni. Detto ciò, questa volta ci aspettavamo un atteggiamento da parte del Governo ben diverso. Ci aspettavamo un'ulteriore fase di ascolto e di confronto, al solo fine di migliorare le norme previste in questo testo e meglio modellarle al mutato contesto di mobilità delle nostre strade. Invece no: siamo di nuovo qui. Il Senato è in seduta a ratificare il lavoro svolto dalla Camera e questo perché e questo perché probabilmente non siete nemmeno in grado di organizzare i lavori parlamentari. Ovviamente non è solo questo il motivo che ci indispone a votare favorevolmente il vostro nuovo codice della strada: c'è ben altro. Devo entrare nel merito anche dopo aver ascoltato gli interventi

Io vedo semplicemente dei parlamentari che rinnegano il loro ruolo di legislatori e giustificano le carenze di questo Governo, anche nel dialogo che dovrebbe essere fatto all'esterno con le persone interessate dal codice. Come dicevo, vado nel merito, anche perché davvero non riuscirei ad esprimere tutto quello che ho da dire su questo codice. I dieci minuti non mi bastano per la dichiarazione di voto e cercherò di essere sintetica. All'articolo 1, sia ben chiaro, a noi sta bene la stretta aggiuntiva che è stata riservata a chi guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e uso di sostanze psicotrope. Peccato che voi non fate solo questo, ma andate ben oltre. ma andate ben oltre. Voi andate a cancellare quella frase «in stato di alterazione psicofisica», che è l'unico elemento che potrebbe garantire la possibilità per un soggetto di provare il contrario. E questo perché oggi sappiamo benissimo che esistono dei medicinali che contengono delle sostanze che, se assunte per settimane, possono produrre una reazione positiva al test che verrebbe loro fatto. Parlo del paracetamolo, o della codeina: si tratta di semplici analgesici, antidolorifici che probabilmente anche noi in quest'Aula utilizziamo quando abbiamo dei dolori, ma che sicuramente persone affette da tumori o da fibromialgia sono costretti ad utilizzare. Allora, con questa modifica al codice voi andate andate a inserire indirettamente un divieto che - sia ben chiaro - siete liberi di fare, ma non nel codice della strada; voi potete indicare un divieto; ponete per legge il divieto di consumare farmaci di questo tipo, il divieto di assumere droghe e non capisco perché non lo fate. Lo fate Lo fate qui dentro, in maniera indiretta, andando a travisare anche quello che la Costituzione ci garantisce. qui ravvedo l'incostituzionalità della norma, proprio per effetto del ragionamento che vi ho fatto, ovvero l'inserimento di un divieto indiretto. Ma questi sono concetti che sono chiari ai medici, ai giuristi, tranne che a voi ovviamente, esattamente come non interessa a voi capire la differenza tra CDB e THC. Che cosa c'entra questo? È molto semplice: perché la questione fa il paio con quello che avete inserito nel disegno di legge sicurezza, che è ancora in discussione qui in Senato, e dove proibite la commercializzazione di prodotti contenenti CDB e non THC, che è cosa ben diversa. è cosa ben diversa. Non so perché davvero non fate un provvedimento dove vietate l'uso di queste sostanze in maniera chiara. Voi ve ne daremo atto e ve lo voteremo pure, perché ad oggi questo non c'è e non esiste. Non so che cosa vi trattenga. Soprassiedo sull'articolo 7 le limitazioni ai neopatentati, perché ne ho già discusso in fase di illustrazione degli emendamenti e vado avanti, continuando sulla vostra spasmodica ricerca del nemico numero uno della sicurezza stradale, che finalmente avete trovato e avete inserito nell'articolo 14. Che bravi! i monopattini elettrici, l'oggetto della discordia, il monopattino elettrico di proprietà privata o in condivisione, in *sharing*, da qualunque punto lo si voglia guardare. Come dimenticare allora le parole della presidente Meloni, che dichiarò nell'ottobre 2022 alla Camera dei deputati: «Non disturbate chi vuole fare». Ma siamo sicuri? Siamo sicuri di chi stiamo parlando? No, perché con targa, casco e assicurazione a me non sembra che voi non stiate disturbando un settore che ad oggi ha raggiunto un fatturato di 119 milioni di euro, che ad oggi ha 2.300 addetti dipendenti, che ad oggi ha 100.000 monopattini sparsi su tutte le strade d'Italia; un settore che, da quando è stato introdotto il monopattino nelle strade, dal 2019 ad oggi, ha raggiunto un incremento del 39 per cento dei noleggi: una crescita spropositata in un ambiente che decresce economicamente. È soprattutto il casco, rendendolo obbligatorio per ogni età, la scure che abbatterà almeno il 70 per cento dell'utilizzo dello *sharing* dei monopattini, con buona pace, Presidente, di chi voleva fare, che stava facendo e che stava facendo pure bene, appunto. E se consideriamo che la contrazione della domanda dello *sharing* si riverserà sul ritorno all'uso dell'auto privata da parte di queste persone, il danno è anche doppio, a causa delle nuove immissioni in aria di CO2 e particelle inquinanti. E arrivo all'articolo 15, quando invece troviamo il grande *bluff*, Ministro, il suo grande *bluff*, con tutta la maggioranza al seguito, ovviamente. Attenzione, però, questo non lo dico io, ma lo dicono centinaia

ad arrivarci *mail* - di rendere dignità ed onore a quelle persone, ai ciclisti morti a causa di una collisione con un'automobile. L'innovazione legislativa che obbliga un automobilista a procedere al sorpasso di un ciclista garantendo la distanza di un metro e mezzo dallo stesso viene completamente svilita dalla frase che la segue, ovvero «ove le condizioni della strada lo consentano». Ci siamo fatti portavoce allora delle istanze di tutti i cittadini che sono qui fuori a dimostrare contro di voi, con soluzioni interpretative della norma per migliorare la definizione dei casi, ma la vostra sordità ha raggiunto veramente dei livelli mai visti. Ma andiamo avanti e lo faccio saltando a piè pari l'obbrobrio delle sanzioni cumulative relative agli autovelox, che non è certo un deterrente alla fretta che fa pigiare sull'acceleratore dell'auto. Piuttosto invece è utile a creare un ambiente giuridico che diventa complesso da gestire da parte dei Comuni, quando devono elevare una multa. Arrivo alle Zone 30 e mi dispiace che il Ministro sia andato via, perché volevo ricordargli un po' le sue azioni. Quelle irragionevoli Città 30, quelle aree di mobilità lenta a cui il Ministro ha promesso una grande battaglia, concentrandosi però solo su un Comune, quello di Bologna, e dimenticando quello di Olbia. Il Comune di Olbia è amministrato da un sindaco che siede nelle fila di Forza Italia sin dalle prime ore; nel 2021 forse è stato proprio lui il pioniere dell'attuazione delle prime Città 30, non solo all'interno della città urbana e del centro urbano, ma anche nelle frazioni. Lui si chiama Nizzi ed è convinto che la Zona 30 sia la via giusta e che Salvini semmai debba imparare a rispettare l'autonomia dei territori. Ma Nizzi non è solo, no, perché ci sono il sindaco di Vicenza, il sindaco di Verona, l'ex sindaco di Genova, il sindaco di Treviso e Salvini stesso, che nel febbraio 2023 ha stanziato ha stanziato ben 13 milioni di euro proprio sulla sicurezza dei pedoni, facendo riferimento all'implementazione delle Zone 30, per mitigare la differenza delle velocità esistenti tra pedoni e traffico motorizzato. Allora, Presidente, mi avvio alla conclusione… Ha parlato anche ieri: le do trenta secondi. DI GIROLAMO *(M5S)*. Va bene, Presidente, chiudo molto velocemente. Noi non ci macchieremo le mani di rosso, di sangue, come state facendo voi. Noi stiamo ascoltando le persone che fuori ci stanno chiedendo di fermarvi, di farvi riflettere,

Presidente, Governo, ovviamente ce ne faremo una ragione se non avremo il voto favorevole dei 5 Stelle, che è solito sempre insultare.

Signor Presidente, oggi con molta soddisfazione intervengo in dichiarazione di voto, a nome del Gruppo Lega, sul disegno di legge presentato dal ministro Salvini, che reca interventi in materia di sicurezza stradale. Prima di procedere, voglio ringraziare il ministro Salvini per il suo straordinario lavoro *(Applausi)* nel portare avanti una riforma tanto necessaria quanto coraggiosa. E rispondo agli attacchi di chi non ha saputo cogliere il valore della nuova legge. Voglio ribadire invece l'importanza della sua determinazione nell'affrontare un tema che incide profondamente sulla vita quotidiana di ogni cittadino. Il ministro Salvini ha dimostrato una visione chiara e una ferma volontà di offrire finalmente un codice della strada organico, ponderato e lungimirante. di una riforma di assoluto buonsenso, pensata per rispondere alle esigenze reali delle comunità - perché noi ci confrontiamo con le comunità, a differenza di chi invece non lo fa e pretende in quest'Aula di strumentalizzare - e per garantire una maggiore sicurezza sulle nostre strade. A differenza di quanto fatto negli anni

con particolare attenzione soprattutto ai giovani e agli utenti più vulnerabili della strada. Le critiche ricevute, che sono strumentali, non intaccano ovviamente la portata di questa riforma che introduce misure concrete per tutelare la vita delle persone e promuovere una cultura del rispetto e della responsabilità sulle nostre strade. È proprio grazie a questa visione strutturata e al lavoro instancabile del ministro Salvini che possiamo guardare con fiducia a un futuro in cui la sicurezza stradale diventi una priorità vera e È nato così un insieme di norme che tocca tutta una serie di aspetti, anche nuovi, relativi alla sicurezza stradale ed elaborati attraverso un'istruttoria molto attenta e articolata che ha tenuto in gran conto i contributi dei gruppi di soggetti interessati. Infatti sono state numerosissime le audizioni Grazie a tutti uscendo da quest'Aula, mi sono imbattuta in alcuni rappresentanti delle associazioni di familiari di vittime della strada, che mi hanno ringraziato e mi hanno chiesto di portare i loro ringraziamenti anche al ministro Salvini per questo codice della strada. Molte delle proposte arrivate da quei gruppi sono state recepite, a riprova di quanto per noi sia importante l'ascolto. Le numerose modifiche apportate al testo iniziale dimostrano l'attenzione con cui questo lavoro è stato condotto, per arrivare a un testo finale il il più possibile condiviso e rispondente alle concrete esigenze della sicurezza dei cittadini. Spiace quindi che i colleghi di opposizione, per mera propaganda politica, si siano scagliati contro questo disegno… *(Commenti).* che prevede interventi volti a garantire una mobilità più sicura per i cittadini. D'altronde la passione - consentitemi di dirlo - con cui il ministro Salvini ha portato avanti questa riforma nasce proprio da una dolorosa constatazione che non consentiva più di rimandare ulteriormente l'intervento. Mi riferisco al numero dei morti sulle strade. Non sto qui a elencare i dati, ma quegli incidenti incidenti sempre più vedono coinvolti monopattini e mezzi di micromobilità elettrica, sempre più utilizzati soprattutto nelle grandi città, dove certamente si dimostrano utilissimi per bypassare il traffico cittadino o comunque per spostamenti rapidi e improvvisi, ma sono sempre più usati in maniera scorretta e selvaggia, con la conseguenza di un numero sempre più crescente di incidenti anche mortali, soprattutto tra i più giovani. Ci dispiace dover disturbare le aziende che affittano i monopattini, che dovranno certamente riorganizzarsi, ma a noi sta a cuore la vita dei cittadini e non certo i fatturati delle aziende. Cause di queste morti sono principalmente la distrazione, l'uso del telefonino alla guida, ma anche l'alta velocità, la guida in stato di ubriachezza o sotto sostanze stupefacenti, cioè la violazione stessa delle norme basilari della sicurezza stradale; soprattutto, tra i ragazzi non ci si rende conto di quanto mettersi al volante, per esempio, dopo aver bevuto possa essere pericoloso per sé e per gli altri. Citando alcuni dati a questo riguardo, provenienti dai Carabinieri e dalla su 52.459 incidenti con lesioni, 5.085, cioè ben il 10 per cento, si sono verificati con almeno uno dei conducenti in stato di ebbrezza e in 1.676 è stato accertato l'uso di stupefacenti. Per questo si è reso necessario intervenire partendo proprio da queste constatazioni, prevedendo misure stringenti di prevenzione e sanzioni che vanno a incidere anche sulle norme penali, ma anche misure deterrenti, come la sospensione breve della patente. Questo perché noi abbiamo attenzione e amore per i giovani, al contrario di quanto è stato riferito Un altro capitolo importante, che si interseca con l'aspetto della prevenzione, è quello della formazione, più che mai fondamentale per andare a incidere sulla cultura, sulla visione e anche sulla preparazione del guidatore, soprattutto per cercare di educare nel tempo a una guida responsabile e attenta, facendo capire quanto una distrazione, anche piccola e semplice, possa essere fatale, e dunque quanto sia indispensabile una responsabilizzazione personale. L'educazione stradale, stradale, che già rientra nei programmi di educazione civica nelle scuole, reintrodotta grazie ad una legge proposta dalla Lega, sarà oggetto anche di corsi extracurriculari per gli studenti delle scuole superiori. Alla formazione, poi, affianchiamo anche un rafforzamento del sistema dei controlli con violazioni accertabili anche da remoto, proprio per scoraggiare comportamenti sbagliati o superficiali; tra questi, anche l'abbandono di animali sulle strade. Per tale ipotesi vengono giustamente inasprite le pene fino a sette anni anni di carcere, sia nel rispetto dei nostri piccoli amici a quattro zampe, che hanno diritto di essere amati e tenuti da chi ne abbia davvero cura, sia per prevenire terribili incidenti causati dagli animali lasciati incivilmente sulle strade dai padroni. Un ultimo punto sul quale vorrei soffermarmi è quello della velocità nei centri urbani. Anche a questo proposito il nuovo codice della strada prevede, sì, pene pesanti con il ritiro immediato della patente quando si superano i limiti di velocità nei centri urbani; tuttavia, riguardo alle Zone 30, che qualcuno ha definito visione di una nuova mobilità sostenibile, noi di certo diciamo sì alle Zone 30 vicino alle scuole, nelle strade dove c'è intenso traffico di pedoni e ciclisti, ma non possiamo acconsentire alle ordinanze ideologiche di chi vorrebbe imporre le Zone 30 in tutte le città, creando solo un disagio ai cittadini, senza alcun beneficio a favore della sicurezza. *(Applausi)*. Credo quindi che il lavoro del Ministro non si sia limitato a rispondere a necessità contingenti o a richieste dettate dall'urgenza del momento, ma abbia mirato a costruire un sistema che mette al centro la tutela della vita, la sicurezza di tutti gli utenti della strada e la prevenzione di comportamenti pericolosi. Questo approccio, tanto strutturato quanto lungimirante, dimostra cosa significa davvero fare politica per il bene del Paese: offrire soluzioni durature, concrete, responsabili e capaci di migliorare la qualità delle persone Grazie a questa visione, il ministro Salvini e la Lega stanno tracciando una strada - per restare in tema - che non solo innova, ma rafforza la fiducia nelle istituzioni, dimostrando che si può e si deve lavorare con determinazione

Signor Presidente, colleghe e colleghi, siamo chiamati - e ne siamo consapevoli - a votare un provvedimento che avremmo voluto rappresentasse davvero una svolta nella tutela della vita umana sulle nostre strade. Così la maggioranza - lo abbiamo ascoltato - continua a ripeterci, ma non è così nei fatti. Il nuovo codice della strada che sta per diventare legge tradisce le aspettative dei cittadini, delle amministrazioni locali e soprattutto delle famiglie che ogni giorno convivono con il dolore di una perdita evitabile. Non possiamo chiudere gli occhi, il testo che abbiamo davanti è un'occasione mancata e in molti aspetti addirittura un passo indietro. Ieri, durante la discussione generale, oggi nel dibattito sugli oltre 300 emendamenti, tutti abbiamo ricordato le tragedie che accadono sulle nostre strade. Venerdì l'Istat ha pubblicato le stime preliminari sugli incidenti stradali in Italia nei primi sei mesi del 2024: tra gennaio e giugno c'è stato un incremento, rispetto allo stesso periodo del 2023, del numero di vittime sia sulle strade urbane (+8 per cento), sia su quelle extraurbane (+1 mentre le stime indicano una diminuzione delle morti in autostrada. Sono dati che dovrebbero preoccupare, soprattutto considerando che le modifiche al codice della strada interverranno in misura maggiore sulle strade urbane ed extraurbane, rendendo più difficile l'utilizzo dei dispositivi di controllo automatico, delle violazioni dei limiti di velocità e limitando limitando la possibilità delle amministrazioni comunali di abbassare invece il limite da 50 a 30 chilometri all'ora. Ogni giorno in Italia muoiono otto persone, oltre 600 rimangono ferite e non sono solo numeri, parliamo di progetti interrotti, di vite spezzate, di famiglie distrutte, sono tragedie che ci chiedono di agire con responsabilità, di avere il coraggio di scegliere misure che invertano questa inaccettabile deriva di morte. Come hanno scritto le associazioni dei familiari delle vittime, si tratta di decidere se volete dare o meno priorità alla protezione della vita. Questo codice purtroppo non lo fa, questo codice ignora i veri problemi. Le cause principali degli incidenti stradali in Italia sono note: eccesso di velocità, distrazione alla guida, mancato rispetto della precedenza. Non lo diciamo noi, lo dicono i dati ufficiali, ma questo testo, invece di affrontarle, sembra minimizzarle, permette ai neopatentati di guidare auto potenti, nonostante siano una delle categorie più vulnerabili; introduce il concetto assurdo delle sanzioni cumulative, per cui un conducente può infrangere ripetutamente i limiti di velocità nell'arco di un'ora ricevendo una sola multa;

miope, anacronistica. In un momento in cui l'Europa guarda al futuro della mobilità sostenendo alternative all'uso dell'auto, questo codice torna indietro, penalizza chi sceglie di muoversi in modo sostenibile, impone obblighi e restrizioni alle biciclette e ai monopattini, equiparandoli ai mezzi motorizzati, come se rappresentassero il problema anziché una parte della soluzione. inoltre, la realizzazione di piste ciclabili e scoraggia l'uso delle bici con norme contraddittorie; rende più difficile l'istituzione di zone a traffico limitato e di aree pedonali, strumenti che non solo migliorano la qualità dell'aria, ma salvano vite. Le città che hanno avuto il coraggio di adottare le Zone 30, come Bologna e non solo, hanno visto una riduzione degli incidenti del 20 per cento. Berlino, con misure simili, ha abbattuto le emissioni di ossidi di azoto del 40 per cento. Questo è il futuro, non si può ignorarlo e, come ha già ricordato ieri la collega Zampa, i cittadini di Bologna lo hanno capito e hanno premiato questa scelta. *(Applausi)*. Questo codice, invece, è calato dall'alto, non ascolta il grido dei cittadini e la voce dei territori. Quando abbiamo audito le associazioni delle famiglie delle vittime -tutte le associazioni - queste ci hanno rivolto un appello chiaro: fermiamo questo testo, riscriviamolo. Sono loro a ricordarci che le strade più sicure non si costruiscono con norme punitive, ma con prevenzione, formazione, tecnologia e responsabilità. Allo stesso modo, i sindaci, che sono i primi a conoscere i bisogni della comunità, sono stati esautorati. Questo codice centralizza decisioni fondamentali, sottraendo ai Comuni la possibilità di istituire ZTL, piste ciclabili, misure per ridurre la velocità, come hanno ben evidenziato nel dibattito i colleghi Irto e Delrio. Come possiamo ignorare la voce di chi vive e amministra i territori, di chi ogni giorno vuole dare risposte ai cittadini che chiedono più sicurezza? Ma non vi rendete conto della follia di voler spaccare l'Italia sulla sanità, l'istruzione e le politiche energetiche e poi voler decidere a Roma, al Ministero, dove posizionare i cartelli stradali e la velocità delle singole rotonde e delle strade urbane? Cerchiamo di capire la valenza e la portata di quello che stiamo decidendo oggi; non stiamo votando solo un testo di legge, stiamo decidendo che tipo di società vogliamo essere, se vogliamo continuare a leggere ogni giorno numeri che somigliano a un bollettino di guerra o se vogliamo impegnarci a costruire strade più sicure, città più vivibili, un futuro più giusto. Oggi questa è la nostra sfida: avere il coraggio di dire no a norme che tradiscono la protezione della vita ed impegnarci per riscriverne di nuove e più tutelanti. Alle famiglie delle vittime va il nostro impegno; le loro voci oggi risuonano in quest'Aula, attraverso i dati, le storie, le richieste di buonsenso che ci hanno presentato e che ha ricordato la collega Floridia. Non possiamo tradire la fiducia di chi ha Non possiamo accettare un codice che, come hanno detto loro stessi, garantisce il perpetuarsi della strage stradale. Se non si investe nella mobilità sostenibile e alternativa all'uso dell'automobile e nella tecnologia, come si intende ridurre il numero di auto in circolazione, la quantità di emissioni, il numero di incidenti?

Grazie a tutti Questo è il futuro della mobilità ed è una battaglia che il Partito Democratico continuerà a portare avanti, specie di fronte alla miopia cronica di questo Governo. Serve però l'impegno di tutti, perché la sicurezza stradale è una battaglia che riguarda ciascuno di noi. Non possiamo più permetterci di aspettare; ogni giorno perso significa altre vite spezzate, altri sogni infranti. Abbiamo il dovere morale e politico di fermare questa strage silenziosa. Noi continueremo a lottare per questi obiettivi in Parlamento e nei territori.

il disegno di legge che oggi stiamo discutendo merita tutta la nostra attenzione. La sicurezza stradale è un tema molto delicato e rappresenta uno dei problemi più gravi della nostra Nazione, che resta uno dei Paesi più motorizzati d'Europa e con elevati livelli di incidentalità. Le statistiche in tal senso sono molto allarmanti. I dati relativi al 2023, che quest'oggi sono stati più volte ricordati, danno un quadro molto preoccupante, 166.000 incidenti, approssimativamente 456 al giorno, causando la morte di oltre 3.000 persone. Ciò significa che otto persone ogni giorno perdono la vita a causa degli incidenti stradali. che nel nostro Paese, che sta invecchiando sempre più, gli incidenti stradali rappresentano la prima causa di morte nella fascia d'età tra i quindici Ho scelto di iniziare questo mio intervento citando queste tragiche statistiche per dare il senso di quanto sia importante e delicata la tematica che stiamo affrontando quest'oggi. Di fronte a questo scenario, la politica non poteva rimanere indifferente e il Governo Meloni ha scelto di non restare a guardare. Era necessario intervenire tempestivamente per fermare queste continue stragi sulle strade italiane che ogni anno spezzano il futuro di tanti connazionali, devastano le famiglie, cancellano sogni, desideri e ambizioni, soprattutto dei nostri giovani. La revisione del codice della strada non rappresenta dunque un documento tecnico composto di regole, istanze e percentuali. La revisione del codice della strada rappresenta la chiara volontà politica di questo Governo di tentare di mettere un freno a questa mattanza di vite umane che insanguina le nostre strade. È un tema che tocca ciascuno di noi; chi guida, chi non ha la patente, chi va in bicicletta, chi semplicemente passeggia. È un tema che riguarda ogni fascia d'età: anziani, adulti, adolescenti e perfino bambini. Pensate che addirittura sono in aumento i decessi a seguito di incidenti nella fascia di età tra zero e quattrodici anni. La revisione del codice era dunque una priorità del Governo Meloni. Non si poteva più aspettare. Era necessario rivedere un testo risalente al 1992, ormai vecchio di trentadue anni, un periodo in cui il mondo della mobilità è notevolmente cambiato. È stato svolto un lungo lavoro e permettetemi oggi di ringraziare il ministro Salvini, il vice ministro Bignami, il sottosegretario Ferrante, che con noi ha condiviso molte ore in Commissione, i relatori e tutti i membri della Commissione.

poiché in una Nazione dove sulle strade muore una persona ogni tre ore era fondamentale approvare il provvedimento il prima possibile. Abbiamo quindi deciso di ritirare tutti i nostri emendamenti, trasformandoli in ordini del giorno vincolanti, affinché possano essere recepiti nell'ampia delega al Governo contenuta nel disegno di legge. Non abbiamo la presunzione di affermare che questo disegno di legge risolva tutti i problemi, ma possiamo sicuramente affermare che questo testo mette finalmente un argine a chi scambia le autovetture per cabine telefoniche, a chi usa le auto come *set* per diventare *youtuber* e a chi scambia le strade per piste di Formula 1. *(Applausi)*. Non siamo disponibili a tollerare chi gioca o scherza sulle nostre strade. Si tratta, dunque, di una normativa volutamente più severa più severa nei confronti di chi guida in stato di ebbrezza. Agli automobilisti condannati per i reati di guida in stato di ebbrezza potranno essere applicate limitazioni alla guida con l'obbligo di installazione del dispositivo di blocco di tipo alcolock, che eviterà l'accensione dell'autovettura nel caso in cui il guidatore abbia un tasso alcolemico superiore allo zero. La normativa è più severa anche nei confronti di chi fa uso di droga. Le Forze di polizia vengono messe nelle condizioni di contestare più facilmente il reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Finalmente si potranno svolgere sul luogo del controllo accertamenti preliminari con test salivari e, in caso di esito positivo, potrà essere direttamente impartito il divieto di proseguire il tragitto. Si afferma quindi il principio fondamentale chi guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti viene punito senza dover verificare lo stato di alterazione derivante dall'assunzione della sostanza. Questa revisione del codice

infatti un pericolo per te e per gli altri e lo Stato non è disponibile a farti sconti. Questo è un codice più severo anche nei confronti di chi usa il telefono alla guida. La distrazione alla guida resta infatti la prima causa di incidenti stradali. Con questo nuovo codice, chi utilizza il telefono alla guida sarà soggetto non solo a una multa più elevata rispetto al passato, ma anche alla sospensione della patente da quindici giorni a due mesi. anche nei confronti di un'altra piaga della nostra Nazione, l'eccesso di velocità, con l'inasprimento delle sanzioni e con la possibilità di sospensione della patente da quindici Il disegno di legge si occupa anche dei monopattini elettrici, il cui uso è aumentato notevolmente negli ultimi anni e purtroppo sono aumentate anche le vittime tra gli utenti di questi mezzi. Finalmente anche questi mezzi dovranno essere dotati di contrassegno identificativo e assicurazione. Chi li guida dovrà indossare un casco e il loro utilizzo sarà consentito solo su strade urbane. Non vedremo più monopattini sfrecciare e correre su piste ciclabili, marciapiedi e aree pedonali. Non si tratta di una guerra contro queste nuove forme di mobilità, ma semplicemente di promuovere un uso consapevole e sicuro di questi mezzi sulle strade. Non si può però parlare di sicurezza stradale senza incentivare e investire nell'educazione e nella cultura della sicurezza. Il provvedimento in approvazione promuove e incentiva la partecipazione a corsi extracurriculari di educazione stradale organizzati dalla scuola. L'obiettivo è che soprattutto i più giovani comprendano quanto sia fondamentale per la salvaguardia della propria e dell'altrui incolumità adottare un comportamento corretto quando si trovano al volante. La revisione del codice introduce norme più severe nei confronti degli incivili che abbandonano gli animali domestici sulle strade, con l'introduzione di pene rafforzate. *(Applausi)*. Questo provvedimento non solo tutela gli animali, ma mira anche a scongiurare i pericoli che potrebbero derivare per gli utenti della strada. Potrei continuare per ore a a raccontare gli elementi qualificanti di questo provvedimento, ma penso che il dibattito e soprattutto gli interventi del centrodestra e di Fratelli d'Italia siamo stati abbondantemente esaustivi. dalle opposizioni dire che questo codice sarebbe un'occasione persa. Io mi domando: se ci sono, ancora oggi, dei problemi non risolti, vorrei tanto sapere, perché non l'avete detto, cosa avete fatto voi quando eravate al Governo? Mi piacerebbe sapere perché non avete messo in pratica tutti i provvedimenti che quest'oggi avete elencato. Cara senatrice Di Girolamo, chi si è macchiato le mani di rosso in passato? Chi poteva fare e non ha fatto? Prima della dichiarazione di voto, desidero esprimere un profondo e sentito ringraziamento a tutti coloro che, ogni giorno, vigilano sul rispetto delle norme. Fratelli d'Italia rivolge la sua gratitudine agli uomini e alle donne in divisa per il loro straordinario lavoro quotidiano, che garantisce la sicurezza dei cittadini.

la finalità fondamentale del disegno di legge n. 1037 consiste nel riconoscimento e nella promozione della mototerapia. Ricordo che il provvedimento è stato trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. La Commissione affari sociali, alla quale era stato assegnato, ha approvato cinque emendamenti riferiti al testo originario, due dei quali presentati in conseguenza di condizioni formulate dalla 5a Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Successivamente in Assemblea non sono stati presentati emendamenti e lo scorso 21 febbraio la Camera dei deputati ha approvato a maggioranza il testo licenziato dalla Commissione. In Senato, il disegno di legge è stato assegnato in sede redigente alla 10a Commissione, la quale ha proceduto a una trattazione accurata anche per mezzo di audizioni. La Commissione ha infine respinto tutti gli emendamenti posti in votazione e ha approvato a maggioranza tutti gli articoli del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Gli obiettivi essenziali del disegno di legge, esplicitati dall'articolo 1 e ai quali ho inizialmente accennato, sono dunque il riconoscimento e la promozione della mototerapia in quanto terapia complementare, atta a rendere più positiva l'esperienza dell'ospedalizzazione, a contribuire al percorso riabilitativo dei pazienti e ad accrescere l'autonomia, il benessere psicofisico e l'inclusione dei bambini, dei ragazzi e degli adulti con disabilità. Ai sensi dell'articolo 2, entro sei mesi dall'entrata in vigore, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro della salute, sentita l'Autorità politica delegata in materia di famiglia, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con l'accordo della Conferenza Stato-Regioni, sono adottate le linee guida in materia, riguardanti in particolare: gli ambiti di applicazione e gli obiettivi dei progetti di mototerapia e i relativi criteri generali di programmazione, attuazione, monitoraggio le modalità di partecipazione e di supervisione allo svolgimento dei progetti di mototerapia da parte del personale medico e sanitario, dei familiari e delle altre figure eventualmente coinvolte; il coinvolgimento degli enti privati operanti nell'ambito della mototerapia; i compiti e le responsabilità dell'operatore motociclistico, i requisiti e le licenze che lo stesso deve possedere, nonché i relativi percorsi formativi; i protocolli di sicurezza e le misure igienico-sanitarie; la tipologia e i requisiti dei motoveicoli e delle attrezzature utilizzabili; le disposizioni finali e transitorie. L'articolo 3 prevede la facoltà per le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di promuovere l'organizzazione di eventi e di progetti di mototerapia, da attuare con il coinvolgimento di enti privati, anche sportivi dilettantistici e del terzo settore, presso strutture ospedaliere, sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, nonché presso altri luoghi all'aperto o al chiuso idonei a garantire la sicurezza e la piena accessibilità da parte delle persone con disabilità. Infine, l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

a tutti i deputati e i senatori che sono intervenuti in un dibattito costruttivo, all'onorevole Panizzut per la proposta di legge e al senatore Berrino per essere stato relatore del provvedimento. Credo che con questo provvedimento noi portiamo un po' di luce in un percorso di cura che deve rispettare sempre il percorso convenzionale. Abbiamo bisogno tutti delle medicine, delle cure, degli ospedali e dei medici, ma è altrettanto importante una dimensione della vita legata all'umanizzazione delle cure e questo passa anche attraverso la capacità delle terapie complementari (come la mototerapia, ma in futuro spero nel riconoscimento di tante altre, come la musicoterapia, la clownterapia, l'arteterapia e tutte quelle che già conosciamo) di dare davvero un sollievo, un'emozione, una luce, una carezza e qualcosa di più a quei bambini che hanno una malattia grave, cronica, degenerativa, oncologica, rara o una disabilità e spesso vivono in contesti ospedalieri dei periodi temporanei o prolungati, anche di isolamento. Grazie a tutti gli operatori e alle famiglie, che si dedicano agli altri e che davvero credono che la dimensione della vita di ogni persona

intervengo sul disegno di legge in esame non senza imbarazzo nella speranza che quest'Assemblea, sebbene all'ultimo momento utile, risparmiare al Paese, alla medicina, alle difficili storie di malattia, l'umiliazione *(Applausi)* di una legge *spot* senza capo né coda, che introduce nell'ordinamento una pratica priva di alcuna evidenza scientifica. *(Applausi)*. Mi riferisco, tramite lei, Presidente, al Governo: non è un percorso di cura, non è una terapia complementare, non esiste alcuna minima evidenza a sostegno della proposta e della promozione della mototerapia. Con questo disegno di legge si spaccia per terapia quel che non lo che non è terapia integrativa, che non è terapia complementare, ma è attività ludica, così come il gioco a scacchi o il gioco con la palla. E, per favore, vestendo i panni della scienziata, vi chiedo la decenza di non contrabbandare un articolo di valore nullo e privo di misure oggettive, pubblicato sullo «European journal of integrative medicine» come il presupposto scientifico per giustificare questa legge. Perché parlo Sono andata a leggere l'articolo, facendolo anche per dare elementi a voi, e scusate se ne approfitto per spiegare come funziona la scienza e cosa sono le pubblicazioni. Nella relazione illustrativa di questa legge ci si riferisce al citato articolo che tratta di malattie oncologiche pediatriche pubblicato sullo «European journal of integrative medicine», rivista che ha un fattore di impatto di 1.3. Il fattore d'impatto - non so se lo sapete - misura quanto la rivista e le sue pubblicazioni sono di riferimento nel campo. Ecco, un punteggio così basso significa che siamo nella totale irrilevanza scientifica. Per avere un termine di paragone la rivista «Science», su cui ho avuto il piacere di pubblicare anche recentemente, ha un *impact factor* di 47, il «New england journal of medicine», che pubblica articoli in ambito clinico oncologico, ha un fattore di impatto di 91.

delle pubblicazioni da parte degli altri studiosi: più un articolo è citato nelle pubblicazioni successive, più vuol dire che quell'articolo è importante. Ci sono pubblicazioni che accumulano, perché citate dagli altri, decine, centinaia, migliaia di citazioni che aumentano di anno in anno.

Eppure sembra fornire aiuto a malati oncologici, e le pubblicazioni e gli studiosi che si occupano di malattie oncologiche, per giunta pediatriche, nel mondo sono migliaia, sono centinaia di migliaia, sono milioni. Nessuno si accorge di nessuno lo cita. Le citazioni sono a zero. Mi correggo: ce n'è una, di citazione, ma da parte degli stessi autori, in una loro pubblicazione successiva. Quindi questo lavoro è irrilevante, nessuno se ne accorge. E trovo inverosimile che a citare questo articolo sia il Parlamento, che non ha gli strumenti per dire cosa è terapia.

Che sia nullo lo dice anche l'impianto metodologico fortemente carente. Infatti, vi ricordo che la ricerca, se vogliamo chiamarla così, è consistita nella somministrazione di un questionario:

dopo una sessione in moto di due ore una volta al mese, avessero o meno dolore e quali fossero le loro emozioni. Lo stesso è stato fatto sui cinquanta genitori che li seguivano e su venticinque professionisti. Quindi, uno schema fragile, trattandosi di un questionario privo di misure oggettive quantitative. Il terzo elemento che dimostra che è nullo è l'assenza dei controlli. Non Non è stato verificato come si comporta un analogo gruppo esposto ad altro intervento o attività. Potrebbe farli sentire ancora meglio giocare agli scacchi o la musicoterapia, per la quale, invece, esistono evidenze del fatto che riduce la necessità di analgesici ed anestetici in interventi pediatrici. *(Applausi)*. Oppure, potrebbe bastare l'attenzione che si dedica a questi bambini oncologici e il fatto di distrarli dalla loro malattia. malattia. Che sia nullo lo dimostra anche l'assenza di un *follow up*, cioè cosa succede il giorno dopo e qual è l'effetto su parametri medici misurabili. Il mio maggiore sconforto, però, deriva dall'osservare come il Parlamento sia costantemente incapace di discernere tra realtà e finzione quando legifera su temi che riguardano innovazione, scienza e medicina; incapace di attrezzarsi metodologicamente per affrancare quello su cui legifera alle migliori conoscenze disponibili. Ovviamente, le attività ludico ricreative e l'attività fisica ed intellettuale, le azioni di stimolo alla curiosità, che quotidianamente si fanno senza bisogno di leggi,

è, davvero pensate che disciplinare con legge questa singola attività, tra le molteplici possibili, sia qualcosa di minimamente sensato?

Non so se lo sapete, ma la mototerapia è fortemente discriminante. Infatti, molti pazienti pediatrici ne sarebbero esclusi. Non sarebbe meglio immaginare, come è stato osservato nel corso dei lavori della 10a Commissione, se intervento parlamentare deve essere, una cornice legislativa unica, demandando a fonti di grado diverso, alla luce delle evidenze validate dall'Istituto superiore di sanità, se si manifesteranno, l'eventuale regolamentazione di queste attività? Visto che le prove a sostegno della mototerapia sono uguali a zero, può qualcuno spiegarmi, qui in quest'Aula, adesso, perché proprio la mototerapia debba essere riconosciuta dalla legge? Qual è il criterio? È forse dimostrato che sia più efficace delle altre attività? Però, dovete dimostrarlo. Colleghe e colleghi, approvando questo disegno di legge, voi scrivete una nuova pagina imbarazzante della legislazione anti scientifica di questa legislatura. Ce ne sono state altre. L'unico riscatto che vedo possibile è avere il coraggio di bocciare questo In questo senso avevo presentato degli emendamenti in Commissione e col medesimo auspicio intervengo oggi, perché ritornare sui propri passi penso sia molto più dignitoso che perseverare in scelte francamente imbarazzanti.

figlio dell'oscurantismo pregalileiano, mi dà la forza di andare avanti. Ormai da tempo non sentivo uno scienziato, o tale definitosi, porre una finestra sul mondo della realtà di persone in crisi di vita come se fosse una verità assoluta: io sono tutta la scienza, gli altri no. È veramente una schifezza. Se permettete, nel mio piccolo, essendo stato oggetto di scienza sbagliata per tanti anni, ma anche, con un minimo di risarcimento narcisistico, presidente dell'Istituto italiano degli affari sociali, il più antico

Peraltro, anch'io ho uno scooter che fa le veci delle mie gambe, non da qualche anno, per un errore medico di pseudoscienziati. Allora, credo che bisogna discutere su quante possibilità offriamo a persone che hanno una ridotta capacità di scelta, soprattutto bambini,

l'immagine diretta, se posso permettermi, ad alto livello, perché ho rappresentato l'Italia nel mondo scientifico nel più antico e se vogliamo glorioso istituto di ricerca pubblico italiano. Io dico questo: perché cercare di distruggere e non valorizzare delle opzioni di libertà? Perché prendiamo persone che hanno realtà di mobilità, di emozioni e

vivere le emozioni che hanno visto tanto spesso in televisione, tanto spesso nei *media*, tanto spesso tra compagni che li superano in velocità, ma non li superano nella capacità di sognare, forse. Io lo dico da antico, vecchio, forse un po' rincoglionito neuropsichiatra infantile: forse dire "no" a questa finestra sul mondo così complicata da vivere, se non attraverso un nostro interessamento, beh sarebbe un atto di crudeltà, sarebbe un atto di oscurantismo, un atto di chiusura per essere puri. Ma cos'è la purezza, ragazzi? Scherziamo? Quante volte l'*impact factor* è condizionato da interessi privatissimi? Nessuno è puro, nessuno è completamente serio in certe realtà; lo dicevano

sempre dalla parte della ragione e voi avete sempre torto"? Questo non è scientifico, questo non è leale, questo non è politico. Allora io dico, con enorme serenità, che è un provvedimento al limite, che cerca di combattere la ipermedicalizzazione, la iperrelazionalità. Uno più uno fa sempre due? No. Qualche volta, Presidente, uno più uno fa tre, perché dobbiamo considerare le emozioni, i sentimenti, le frustrazioni di chi ha poca, pochissima libertà di scelta. Voi la state limitando per pregiudizi, perché, se l'avesse

Qualcuno sarà illuso (ma quante terapie illudono?), ma qualcuno sarà vincente, almeno per un'ora della sua vita quotidiana. Allora io credo una grande responsabilità, perché mi sono preso l'onere di aprire i lavori su un argomento complesso. Ho detto "sì", perché mi piglio l'incarico di essere scomodo, ma di rappresentare sentimenti, emozioni, frustrazioni, la realtà limitata di persone che hanno problemi enormi, che non possiamo restringere nella cornice della cosiddetta scientificità, che nessuno ha mai dimostrato che cos'è veramente. Allora io non promuovo, Presidente, una *deregulation* della scienza. Mi pongo al servizio dell'opposizione per discutere anche fuori dall'Aula, ma sono contento, anche perché certo ostracismo di maniera fa veramente un pochettino arrossire le gote di chi rappresenta l'opposizione. La scienza non è sempre perfetta; al nuovo, deve essere aperta a stimoli, sempre considerando con rispetto immenso l'utente di riferimento, che in questo caso sono, Ministro, sinceramente, persone con enormi difficoltà difficoltà di vita, con enormi limitazioni, che (perché no?) una volta tanto andare in moto farà sentire più libere. Ma vi sembra poco? Possiamo dire di no? Io no!

su una univocità di scienza; che cos'è una ricerca scientifica lo dicono i testi, non lo dice l'opinione, che può essere confutata. Infatti in questo caso non siamo di fronte ad una ricerca scientifica, perché banalmente

molto pesanti, diremmo che la libertà è la cosa più bella del mondo. La moto da sempre, insieme ad altre cose - ad esempio, a me piacerebbe andare a cavallo, cosa che non so fare -,

che verrà indicato un elemento finanziario, altrimenti non ha senso. Si vuol dire che chi ha la moto farà la mototerapia e che chi non ce l'ha andrà in bicicletta? Non credo. Quindi vorrà dire che verranno sottratte risorse da altre parti.

esempio la clownterapia, che viene fatta dai volontari per donare un sorriso (quindi siamo nella fase di donare un sorriso a un bambino). Tra l'altro, è una ricerca fatta sulla mia città, Torino, con cinquanta bambini che non ha avuto eco in altre città, in altri posti, con altri questionari e, come diceva giustamente la senatrice Cattaneo, senza un confronto con altre terapie e senza una indicazione medica veritiera. che in questo caso siamo di fronte a un'associazione di cui fa parte qualche amico - forse gli interessi privati di cui si diceva prima - e a una proposta di legge che è stata presentata per ringraziare un'associazione. Tutto qui. Non siamo di fronte alla scienza, ma di fronte a degli amici che andavano premiati con una legge. *(Applausi).* Abbiamo quindi il Parlamento al servizio dell'amichettismo.

perché: ci sono delle persone malate, dei bambini malati che hanno delle emozioni ed hanno voglia di vivere,

Grazie a tutti

ma noi siamo il Parlamento e dobbiamo fare distinzione tra essere pelosi ed essere scientifici. *(Applausi)*. Siamo il Parlamento, non siamo la parrocchia, non siamo un'associazione caritatevole. Ripeto, siamo il Parlamento, spiace che questo Parlamento effettivamente non capisca la differenza tra cosa vuol dire normare e cosa vuol dire fare della finta carità pietosa.

potrei anche smetterla qui e fare mio (ovviamente non sono capace e non ho nessuna competenza) quello che diceva la senatrice Cattaneo nel suo intervento, in cui ha spiegato benissimo che non c'entra niente niente dal punto di vista terapeutico e scientifico. Non c'è niente di scientifico in questo provvedimento e questo era chiaro anche in Commissione, tant'è che anche alcuni componenti della maggioranza avevano dei dubbi, perché è inutile girarci intorno. Hanno avuto forti dubbi anche alcuni componenti della maggioranza, però, caparbiamente lei, signora Ministra, ha voluto questo provvedimento, questo è il dato vero.

con la musicoterapia, con i *clown,* con il disegno, con ogni cosa che può venire in mente; una persona che, per esempio, non cammina, la si mette su un cavallo e la si fa camminare su un cavallo e, tutto contento ovviamente, si solleva dalla propria condizione; oppure, se uno fa fatica sempre a camminare, va in una vasca e nuota, certamente si sente sollevato. Potrei fare migliaia esempi concreti, che succedono ogni giorno.

diverso, signora Ministra, se si pensasse ad una cornice per una serie di supporti che molto spesso sono dati da associazioni di volontari. L'intervento dei volontari in una situazione di difficoltà non è una terapia, non è un modo di dare sollievo alle persone,

Ma questo è ciò che succede in ogni famiglia normale tutti i giorni, perché questo è il dato e noi facciamo una legge. Una legge per chi, per un'associazione? Ma chi l'ha detto? Per quale ragione? In questo caso si dice che si fa una legge che non ha costi, ma allora che senso ha? Se non ha costi mettiamo tutti, facciamo una discussione diversa su cos'è l'intervento di l'intervento di sollievo, di partecipazione, di contribuzione per le persone che hanno una difficoltà. Questa è la cosa che non si capisce e quindi siamo legittimati, almeno io lo sono, a pensare che ci sia dietro un rapporto

Francamente la cosa migliore sarebbe, se aveste il coraggio, un sussulto d'orgoglio e ritiraste questo provvedimento,

Per noi è impossibile votare un disegno di questa natura, pur condividendo il fatto che una serie di atti serve per

tra le molte lodevoli iniziative parlamentari, esaminiamo oggi un tema di particolare sensibilità, una proposta che prevede il riconoscimento e la promozione della mototerapia. Si intende ora promuovere la mototerapia come terapia complementare, con l'intento di rendere più agevole il percorso di riabilitazione. Essendo una metodologia di riabilitazione per i bambini e per i ragazzi affetti da disturbi del neurosviluppo, la mototerapia diventa uno strumento in più da affiancare alle terapie che si utilizzano per i giovani con disabilità. In Italia 13 bambini su 1.000 sono colpiti da disturbo dello spettro autistico. Grazie alla mototerapia, si possono coinvolgere concretamente i giovani, utilizzando la motocicletta come attivatore emozionale. Allo stesso tempo, vengono attivati l'apparato sensoriale, quello motorio e quello cognitivo, semplicemente coinvolgendo i giovani in quello che da loro è percepito come un gioco di grandi dimensioni. Ormai sono circa vent'anni che la mototerapia viene utilizzata in progetti riabilitativi che coinvolgono i ragazzi in un momento in cui hanno la possibilità di relazionarsi con gli altri. Certamente la mototerapia può essere utilizzata anche con ragazzi che presentano altri disturbi dello sviluppo, ma anche ritardi mentali o psicomotori. È documentato che l'utilizzo della mototerapia attenua i sintomi della malattia; allo stesso tempo i processi con cui

diversive rispetto alle terapie, perché la scienza a volte non va a braccetto con le emozioni umane che possono rappresentare le altre attività. Con questo, dichiaro il voto favorevole dei senatori di Forza Italia.

Che cos'è la mototerapia? Il termine è ingannevole. Mototerapia: ci stiamo muovendo? Facciamo qualcosa? È una terapia con il moto?

Abbiamo chiarito che si tratta di *motocross* e, quindi, di un'attività spettacolare ludica. Vi dirò però una cosa di più. Dalle audizioni è emerso che la parola mototerapia è una proprietà intellettuale e industriale registrata al Ministero dello sviluppo economico, Ufficio marchi e brevetti, approvata in data luglio 2020.

c'è un articolo e c'è una registrazione, sorgeranno dei problemi anche da un punto di vista del marchio che è stato registrato al Ministero dello sviluppo economico.

mototerapia, dice che non ha ancora raggiunto il numero minimo di casi trattati utili a realizzare un articolo scientifico per validarne i dati. E lo dice chi fa la terapia con la moto e non Vanni Oddera, che è campione di motocross. Ma cosa state approvando in quest'Aula? Signor Ministro, questa è una "marchietta"!

Vi invito a prendere in considerazione, ovviamente, non solo l'intenzione. *(Commenti)*. Credo di poter parlare più serenamente con voi se mi lasciate parlare. parlare. In primo luogo, è fondamentale sottolineare come il termine terapia sia strettamente legato a trattamenti medici, comprovati e supportati da solide evidenze scientifiche. Qui non ci sono evidenze scientifiche, ma non solo. Nel corso delle audizioni che abbiamo svolto - vi invito veramente ad ascoltarle anche dopo, quando avrete approvato il provvedimento e vi sentirete in colpa per quello che avete fatto

La comunità scientifica - come ha detto la professoressa senatrice a vita Cattaneo - richiede prove rigorose e validate per raccomandare qualsiasi forma terapeutica, l'importanza di adottare un approccio *evidence based* che vada al di là delle esperienze aneddotiche, e questa è un'esperienza aneddotica. Sapete perché è un'esperienza aneddotica? Lo dico per farvelo capire, perché le parole della professoressa Cattaneo forse non vi hanno colpito profondamente.

un altro aspetto centrale che nessuno qui ha trattato, neanche i miei colleghi, e che merita un'attenta riflessione. Mi riferisco alla mancanza di un disegno di legge quadro che regoli in modo organico le terapie complementari. È questo il vero problema, signor Ministro, e gliel'ho detto anche in Commissione. *(Applausi)*. Senza un'adeguata cornice normativa, il riconoscimento della mototerapia rischia di risultare inadeguato e incompleto, poiché le terapie complementari sono molteplici. E tutti sappiamo quali sono le terapie complementari: la musicoterapia, l'arte terapia e anche quella che lei ha citato in Commissione, la montagna terapia. noi non l'approveremo. Oggi noi approviamo la *freestyle motocross* terapia: questo stiamo approvando. *(Applausi)*. Ebbene, il rafforzamento di uno specifico intervento come la mototerapia senza un regolamento generale per tutte le altre terapie non convenzionali è un errore pacchiano, vistoso e grossolano. *(Applausi).* Questa legge, se approvata, crea una gerarchia di valori tra le varie tipologie di trattamento senza una base giuridica solida su cui fondare tale distinzione. Questo disegno di legge si presenta come una scappatoia per l'approvazione di una pratica senza un quadro normativo chiaro e coerente rispetto a tutte le altre terapie complementari. In Italia, la mancanza di questa disciplina è un problema serio, al quale dobbiamo noi rimediare con una legge quadro. Chi oggi approva questa legge senza la cornice di una legge sulle terapie complementari e integrative è un irresponsabile. Voi tutti siete degli irresponsabili! Non possiamo permetterci di aprire la porta a una segregazione legislativa che rischia di danneggiare l'intero settore Quando avremo approvato questo provvedimento, con queste caratteristiche, in questo modo, con questi articoli, avremo condizionato l'approvazione di tutte le altre terapie complementari. Signor Ministro, non solo è un errore, ma è un

non esistono delle linee guida. Noi andremo ad approvare un progetto di legge, che chiameremo terapia con la moto piuttosto che mototerapia - ma sempre di *motocross* terapia stiamo parlando - senza preesistenti linee guida. È come costruire un edificio senza fondamenta. Ma vi rendete conto di quello che state facendo? Le linee guida dovrebbero essere adottate solo dopo un'approfondita analisi e validazione scientifica. Non si approva un disegno di legge sulla mototerapia e si demanda a dopo l'approvazione delle linee guida. Ma cosa state costruendo? Non possiamo ignorare che stiamo colmando un vuoto legislativo senza avere esaminato a fondo le terapie complementari, le quali richiedono una certezza che questo disegno di legge non fornisce. Questo crea un altro *vulnus*, che è la disparità di accesso. Sapete perché la disparità di accesso? Non entrerà nei LEA, perché è a costo zero e, non entrando nei LEA, chi la potrà fare la mototerapia col *motocross* negli ospedali? Chi la potrà fare? Quanti sono i terapisti che fanno la mototerapia? Quanti e in quante Regioni? E non essendo esigibile, perché non è inserito nei LEA, nei livelli essenziali di assistenza, mi dite le mamme e i bambini che vorranno praticare la mototerapia quando e dove la praticheranno? In Sicilia, in Valle d'Aosta? Dove? Questo creerà disparità di accesso.

Non si può demandare a una successiva analisi l'approvazione. Ma voi sapete che cosa avete scritto? Almeno spero che ve lo siate letto. Chi la farà la mototerapia? Avete letto l'articolo 2? Avete letto chi materialmente farà la mototerapia negli ospedali? La fanno enti privati, anche sportivi, dilettantistici che operano nell'ambito della mototerapia. Chiameremo delle associazioni, che sono degli enti privati, a fare la *motocross* terapia ai bambini. Comunque, Comunque, dopo due anni, non credevo di poter assistere alla vergognosa presentazione di una terapia di *motocross* da dare ai bambini, semplicemente perché dobbiamo soddisfare il ministro Locatelli. Mi scusi, Ministro, lei

uscite dall'Aula. Questa è un'Aula sacra. Uscite da quest'Aula e andate in bagno. *(Applausi)*. Fate qualcosa, per favore. Fate quello che volete, ma dovete uscire. Fatevi un giro in moto. Andatevi a fare un giro in moto *(Applausi)*. Il MoVimento 5 Stelle è contrario e sarà sempre contrario ad atteggiamenti antiscientifici come questo.

in sede di dichiarazione di voto, a nome del Gruppo, nell'annunciare il nostro voto favorevole, vorrei accompagnarla con una riflessione che mi auguro possa aiutarci a vederla in prospettiva. Proviamo a immaginare che non possa essere solo la scienza a portare sviluppo e innovazione nella cura, nel prendersi cura della persona nella sua globalità. La ricerca, infatti, si fa anche provando a combinare elementi che fino a quel momento nessuno ha mai provato ad accostare, oppure a dividerli, andando oltre le certezze scientifiche consolidate, perché un tempo c'era chi pensava che l'atomo fosse indivisibile e poi è arrivato il CERN. Non voglio certo far assurgere a ricerca scientifica la cosiddetta mototerapia *(Brusio. è importante, in una strategia di *welfare* evoluto ed integrato, dare a chi è svantaggiato tutte le opportunità per stimolare capacità e abilità residue, in particolare ad interagire con il prossimo. Qui sì che potranno entrare in giuoco scienziati osservazionali, che dai comportamenti potrebbero trarre spunti per ricerche dalle reazioni dei pazienti. Forse non sarà una "terapia" che porterà qualcuno al Nobel, ma potrebbe essere un supporto per individuare altri metodi da applicare all'utenza eleggibile e quindi da valutare per la tutela delle fragilità, soprattutto pediatriche. Ragion per cui io, che non ho mai voluto neanche un "Ciao", ma ho avuto fratelli che per la moto erano disponibili alla qualunque, ritengo che sia un'emozione che possa far vedere loro e manifestare qualche reazione proattiva e soprattutto far sì che gli osservatori possano comprendere, dai loro gesti e dalle loro reazioni, che strada intraprendere per riabilitarli in modo più apprezzabile. Per queste ragioni, riteniamo che il provvedimento possa essere approvato a invarianza finanziaria e che, qualora, come auspichiamo, in linea con coloro che per primi l'hanno praticata, dovesse consolidare gli esiti delle sperimentalità intercorse, si possa andare a consolidare in questa prospettiva una logica utile ad assurgere a terapia complementare ad ogni conseguente effetto.

sui principi e sugli obiettivi che compongono la proposta che oggi stiamo discutendo. Dalle audizioni agli emendamenti che, come Gruppo Partito Democratico, abbiamo cercato di mettere in evidenza nella discussione,

Non ce l'ho con chi ha portato all'ospedale Gaslini della mia città sicuramente un bel momento e una bella esperienza per quei bambini. Mi riferisco al campione di *motocross* Vanni Oddera, che da bambino tra l'altro amava più i boschi che la scuola. Ma, quando parliamo di terapia e quindi di cura, parliamo di qualcosa di molto diverso, come ci ha ricordato con grande precisione e con grande efficacia la collega senatrice Cattaneo ha bisogno di sperimentazioni, di vidimazioni, di controlli e di monitoraggi. Ma di cosa stiamo parlando? C'è una cosa che mi ha colpito sin da subito. Quando parliamo della mototerapia negli ospedali dei bambini e delle bambine, la stessa senatrice ha fatto un passaggio molto importante: quali bambini possiamo riferirci? Se la mototerapia è un supporto psicologico rivolto innanzitutto ai bambini di lunga degenza, ai bambini con patologie ematologiche (leucemia, aplasia) e ai bambini con patologie oncologiche

devono tagliarsi cortissimi le unghie e anche i capelli. Io per due anni sono entrata rapata in quei reparti perché ogni centimetro, ogni millimetro della propria pelle e dei propri capelli può portare un microbo, che per bambini immunodepressi può anche significare l'aggravamento della patologia e magari anche la morte.

un tentativo - lo ricordava il senatore Mazzella prima - con grande efficacia e anche grande puntigliosità

È una vergogna tutto questo e non può essere sopportato in un'Aula parlamentare. *(Applausi)*. Fermatevi in queste cose, perché così non diamo risposte termini di sostegno psicologico di cui tutti, quando siamo in ospedale, abbiamo bisogno, ma in modo particolare i bambini e le bambine, attraverso le tante iniziative di volontari del terzo settore, non solo di personale medico, che offrono la loro opera.

colpisce le persone e che nelle Aule parlamentari deve essere trattato con rispetto e conoscenza. Il nostro è quindi un convinto voto contrario.

favorire il benessere psicofisico e migliorare l'esperienza di ospedalizzazione di persone con gravi patologie, in particolare in età pediatrica. La mototerapia quale terapia complementare rappresenta una sintesi fra innovazione, solidarietà e attenzione alle persone più vulnerabili; un progetto che racconta come sport e inclusione possano generare impatti concreti sulla qualità della vita. Se è del tutto evidente che non si tratta di una terapia in grado di guarire da una patologia grave, è altrettanto chiaro che possa incidere sulla qualità emotiva con cui i piccoli pazienti affrontano la malattia. I dati raccolti dall'*équipe* medica in uno studio svolto presso il reparto di oncologia pediatrica dell'Ospedale Regina Margherita di Torino hanno evidenziato infatti risultati positivi. I bambini coinvolti hanno mostrato una riduzione nella percezione del dolore, accompagnata da un aumento delle emozioni positive. Anche i loro genitori, spesso travolti dallo stress causato dalla malattia dei figli, hanno riportato un miglioramento del proprio stato emotivo. Lo abbiamo sentito nelle audizioni svolte in Commissione e dalle esperienze che sono state raccontate. È evidente che un intervento del genere non solo tocca le vite di chi soffre, ma offre sollievo alle famiglie. Oggi non stiamo semplicemente discutendo di una terapia complementare, ma stiamo parlando di restituire momenti di gioia e possibilità di inclusione a chi vive situazioni difficili. Le esperienze della clownterapia, della pet-terapia, dell'ippoterapia e della musicoterapia - ne cito solo alcune - hanno già da tempo evidenziato l'importanza delle terapie complementari per migliorare il benessere dei pazienti, influendo sullo stato d'animo di chi è costretto a lunghi periodi in ospedale, riuscendo, con l'interazione giocosa e allegra, a trasformare le emozioni negative di chi vive un disagio sanitario o sociale in emozioni positive. Lo sanno bene i tanti volontari che entrano nelle nostre corsie per leggere una favola e portare doni e giochi, quei supereroi che si calano dai tetti degli ospedali per entrare nelle corsie e strappare un sorriso e un abbraccio, rendendo realtà il sogno di tanti bambini malati e riempiendo di gratitudine il cuore di tanti genitori. Il disegno di legge richiama gli articoli 2 e 3 della nostra Costituzione e il dovere di garantire a tutti i cittadini, in particolare ai più fragili, le condizioni per il pieno sviluppo della propria personalità umana, gli articoli 25 e 26 della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità. *(Applausi)*. Noi confermiamo con convinzione il nostro impegno per perseguire quegli obiettivi richiamati, garantendo l'accesso ad esperienze che possano migliorare la loro qualità della vita. È ovvio che tutto questo deve avvenire e avverrà sempre con il supporto, la supervisione e il coinvolgimento diretto del personale sanitario. legge in esame rappresenta, quindi, un esempio di politiche inclusive che valorizzano la partecipazione attiva di tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro condizioni di salute, per offrire un'esperienza che abbatte barriere fisiche, sociali e culturali. Per queste ragioni, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia.

l'introduzione dello sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e di formazione professionale, di cui la 7a ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi

Presidente, onorevoli senatrici, onorevoli senatori, è oggi all'esame dell'Assemblea il disegno di legge n. 845, riguardante l'introduzione dello sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e di formazione professionale, di cui la 7a Commissione, di cui faccio parte, ha concluso l'esame in sede redigente lo scorso 1° ottobre. Il disegno di legge, a prima firma dell'onorevole Lupi, era già stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

e relazionali, capacità comportamentali, caratteristiche psicologiche, come l'ottimismo, e sistemi motivazionali. Gli studi in materia hanno evidenziato che le competenze non cognitive rappresentano un fattore chiave per la riuscita delle persone nelle diverse dimensioni della vita, dal successo scolastico alla realizzazione professionale, alla stabilità economica, fino alla salute fisica e mentale. La maturazione delle competenze non cognitive, che inizia nei primi anni di vita del bambino, continua nel percorso scolastico e prosegue senza interrompersi per tutta la vita adulta, può essere sviluppata mediante opportuni programmi di carattere educativo. Il disegno di legge al nostro esame - per cercare di velocizzare i lavori, visto che ci sono anche degli impegni che alcuni Gruppi hanno preso con la Presidenza - regolamenta

nella precedente legislatura e, come ha sottolineato il collega Romeo, ha avuto una gestazione abbastanza lunga. Credo però che vada dato merito ai colleghi, onorevoli Lupi e Alessandro Colucci di averlo

Intergruppo ha il pregio, da un lato, della trasversalità e, dall'altro, di avere sempre riconosciuto un ruolo centrale al tema dell'istruzione, dell'educazione e della formazione dei nostri giovani. Si tratta di un provvedimento che riprende come base teorica gli studi condotti in materia dal professor James Heckman, docente dell'Università di Chicago e premio Nobel dell'economia. credo, però, che dobbiamo un ringraziamento speciale anche a tre italiani: Giorgio Vittadini, Giorgio Chiosso ed Anna Maria Poggi, che hanno curato il volume "Viaggio nelle character skills. Persone, relazioni e valori". A loro tre va un ringraziamento speciale, perché conoscono la scuola italiana. I contenuti di questa proposta nascono sui banchi di scuola e nascono dall'esperienza di tanti insegnanti, ai quali, come genitori, dobbiamo tutti un grande plauso per il lavoro che svolgono all'interno della scuola italiana. Ma cosa sono le competenze non cognitive? Si tratta di competenze sociali e relazionali, che aiutano lo sviluppo della personalità e anche del talento dei nostri giovani. Penso, per esempio, all'empatia, alla motivazione, alla creatività, alla capacità di gestire lo stress, ma anche alla proattività e al gioco di squadra. Noi, attraverso lo sviluppo di queste abilità umane e sociali, vogliamo favorire lo sviluppo integrale della persona con l'obiettivo di abbattere la dispersione scolastica, almeno in parte, di superare le diseguaglianze e la povertà educativa, ma anche di favorire lo sviluppo del carattere e della personalità di giovani che non sono meno competenti o meno capaci di altri, ma che, a volte, hanno delle difficoltà di apprendimento legate più a delle questioni interiori non risolte. Pensiamo anche ai NEET, cioè alle persone che non lavorano e non studiano, che in Italia rappresentano il 16 per cento della popolazione, ben al di sopra della media UE, che è dell'11 per cento. Insomma, siamo di fronte ad un cambiamento d'epoca, rispetto al quale anche il sistema della formazione si deve adeguare e trovare nuovi metodi e nuovo slancio. Questa proposta di legge suggerisce tre cose. La prima è quella di fare tesoro e mettere a meccanismo comune di conoscenza i progetti pilota che già esistono all'interno delle scuole italiane. Partiamo dalle buone pratiche e dai risultati che sono stati ottenuti attraverso lo sviluppo delle competenze non cognitive e proviamo a fare un salto un salto di qualità, rendendo ordinamentale quel processo. Il secondo punto è la formazione dei docenti. Io credo che, sviluppando la motivazione,

solo all'acquisizione delle competenze, ma anche allo sviluppo della persona, noi costruiremo il Paese di domani e quindi favoriremo la crescita dei nostri ragazzi. Io penso che sia sicuramente un passo nella giusta direzione. Chiudo, però, dicendo che, per favorire l'ottenimento di questo risultato e il miglioramento degli apprendimenti, è fondamentale ricostruire un'alleanza tra gli studenti, gli insegnanti e le famiglie. Qualche volta noi genitori commettiamo l'errore di giustificare un insuccesso scolastico e di schierarci dalla parte dei nostri figli, piuttosto che favorire un'alleanza con gli insegnanti. Così facendo, non facciamo il loro bene. C'è bisogno di rafforzare, invece, la fiducia, la stima e l'autorevolezza degli insegnanti. Questo dipende anche da come noi genitori intendiamo agire. questa proposta di legge sia un passo nella giusta direzione e un aiuto alla crescita di tutti i nostri ragazzi. Per questa ragione il Gruppo Noi Moderati voterà a favore. Signora Presidente, oggi voglio parlare di un tema che tocca da vicino il futuro dei nostri giovani, la salute della nostra società: la dispersione scolastica e la necessità di integrare le competenze non cognitive nel nostro sistema educativo. Viviamo in un'epoca complessa, in cui i ragazzi affrontano sfide senza precedenti: l'ansia, la pressione sociale, l'isolamento e la competizione sono solo alcune delle difficoltà che caratterizzano la loro quotidianità. Molti di loro si sentono sopraffatti, confusi, privi di motivazione e questo può portare ad un abbandono del percorso scolastico. La dispersione scolastica non è solo un problema individuale, ma è un problema che riguarda l'intera comunità e il nostro futuro collettivo. È qui che entra in gioco la proposta di legge per la prevenzione della dispersione scolastica, attraverso l'introduzione delle competenze non cognitive nel metodo didattico. Cosa intendiamo con competenze non cognitive? Si tratta di abilità umane e sociali che non si legano direttamente al sapere teorico, ma che sono essenziali per lo sviluppo integrale dell'individuo. Pensiamo alla gestione dello stress, all'empatia, al *problem solving*, alla motivazione, alla proattività: queste competenze, al pari delle competenze trasversali, sono cruciali per aiutare i ragazzi a navigare tra le difficoltà della vita quotidiana, a costruire relazioni significative, a trovare il loro posto nel mondo e prepararli ad affrontare le sfide della vita sia dentro, che fuori il contesto scolastico. scolastico. Immaginate un ambiente scolastico in cui non si insegna solo a memorizzare nozioni, ma si forma un individuo capace di affrontare le sfide con resilienza. La proposta di legge, seppure in via sperimentale, mira a integrare queste competenze nelle attività educative, perché vogliamo che ogni studente si senta non solo preparato dal punto di vista accademico, ma anche sicuro di sé, motivato e pronto a prendere decisioni consapevoli. Il Ministero dell'istruzione e del merito, quindi, avrà il compito di sviluppare linee guida chiare per implementare queste competenze, affinché le scuole diventino luoghi di apprendimento, dove i ragazzi possano crescere non solo come studenti, ma come persone. Sarà quindi fondamentale mappare le esigenze già esistenti nelle scuole per apprendere da ciò che ha funzionato e costruire su queste basi. Inoltre, entro pochi mesi dall'entrata in vigore della legge, avremo a disposizione un piano straordinario di azioni formative per i docenti. È essenziale che i nostri insegnanti siano preparati e anche supportati in questo cambiamento. Dobbiamo garantire che siano equipaggiati per affrontare le necessità emotive e sociali dei loro studenti, creando un ambiente inclusivo e accogliente. I nostri insegnanti sono il cuore della nostra istruzione e meritano di essere supportati in questo cambiamento fondamentale. Dobbiamo ricordare che dietro ogni numero di dispersione scolastica c'è una storia, un giovane che per vari motivi si sente escluso o incapace di continuare e non possiamo permetterci di lasciare indietro nessuno. Ogni ragazzo merita di essere ascoltato, supportato e guidato verso un futuro luminoso. Sostenere questo disegno di legge significa investire nel futuro della nostra società e dare a ogni giovane l'opportunità di brillare, superare le difficoltà, costruire un percorso di vita ricco e soddisfacente. Significa costruire una società in cui ogni giovane possa realizzare il proprio potenziale, contribuendo così a un futuro migliore per tutti noi. In conclusione, insieme possiamo fare la differenza nella vita dei nostri ragazzi e contribuire a creare un sistema educativo che non solo insegna, ma forma i cittadini del futuro, pronti ad affrontare le sfide del mondo moderno. Per questi motivi, il Gruppo Forza Italia voterà a favore di questa proposta. Presidente, approfitto dei minuti che mi restano perché, parlando di ragazzi, non posso non fare un accenno alla Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che ricorre proprio oggi. Il pensiero non può che andare a tutti i bambini ai quali le guerre e l'orrore hanno strappato il diritto alla spensieratezza, bimbi costretti a lottare per la vita, anziché giocare con i loro coetanei. Ma anche nel nostro Paese ci sono ancora troppi bambini che vivono situazioni di degrado e povertà. È dovere delle istituzioni mettere in campo ogni sforzo possibile per restituire ai bambini e ai ragazzi il diritto a un'infanzia e a un'adolescenza serene, combattendo ogni forma di disagio e di discriminazione, per far sì che possano sentirsi rispettati, ascoltati e soprattutto protetti. Questo è davvero, credo, il primo obiettivo di un Paese che voglia dirsi civile.

un apprezzamento, perché è da celebrare il fatto che questo provvedimento di legge arrivi in Aula nello stesso giorno in cui si celebra la Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Mi sembra un bel modo

sanciti. Questo disegno di legge sicuramente costituisce una forma, ancorché embrionale (mi sia consentito dirlo), di attuazione

certe volte prendono consistenza in modo diverso dal mero studio accademico. Tutti noi abbiamo conosciuto dei compagni di scuola che magari erano geniali nella loro vita e nella loro espressione, ma poi a scuola avevano un rendimento carente o addirittura tendevano a non frequentare la scuola, perché in quella scuola non si riconoscevano, non si sentivano valorizzati, e apprezzati e venivano isolati, forse neanche compresi. C'è uno studio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza del 2022 (quindi molto recente), che pone in evidenza uno stretto collegamento tra il mancato sviluppo dell'apprezzamento, da parte della scuola, delle capacità non cognitive e trasversali e la dispersione scolastica, cioè dimostra apertamente e direi anche in maniera tecnica come il fatto di non tener conto di queste capacità, che pure esistono e che sono all'evidenza dei professori e dei docenti, porti poi questi studenti ad abbandonare gli studi

La necessità di tener conto delle capacità non cognitive e trasversali è sicuramente cogente, urgente e da prendere in considerazione e valorizzare, dando gli strumenti alla scuola. Riconosciamo che, dietro tanti progetti e tanta buona volontà del corpo docente di voler tenere conto di queste capacità e queste attitudini, c'è una non corrispondenza dei mezzi tecnici e degli strumenti valutativi. Quindi c'è la predisposizione da parte del docente a tenere in considerazione determinate capacità, senza poterle però poi tramutare in un voto o in un apprezzamento accademico, quindi senza poterne tenere conto nei giudizi formali che vengono espressi nella valutazione dei discenti. Da questo punto di vista, che proprio oggi si discuta questo disegno di legge è sicuramente testimonianza dell'impegno da parte del Parlamento

Dico "scolastico" e "formativo" perché, correttamente, questo provvedimento si rivolge non soltanto alla scuola obbligatoria, ma anche ai percorsi di formazione professionale e ai CPIA, quindi anche agli studenti adulti, che sono una grande fetta della popolazione, i quali, per vari motivi, non hanno potuto studiare nell'età scolare, magari perché non apprezzati o perché non sono stati messi in condizione di poter coltivare il loro diritto allo studio e che da adulti invece dimostrano la volontà di voler recuperare. Quindi ben venga, da questo punto di vista, un disegno di legge che si incarica di tener conto di queste specificità, di valorizzarle e di trasformarle in percorsi formativi, dando gli strumenti al personale docente per poterli docente per poterli sviluppare, valutare e tradurre in linee guida che potranno essere estese a tutto il comparto scolastico dell'istruzione.

di formazione e di valutazione. Da questo punto di vista, l'apprezzamento verso il disegno di legge in discussione è assolutamente sincero, perché c'è bisogno di apprezzare queste capacità e queste competenze non cognitive e trasversali. C'è un ulteriore tema che va sviluppato e approfondito, ed è quello relativo ai drammi che si sono verificati tra i nostri ragazzi dopo il Covid, con lo sviluppo di disturbi alimentari in percentuale elevatissima (quasi il 60 per cento nella fascia tra i quindici e i diciannove anni). Perché faccio riferimento al Covid? Perché il Covid, causando la sospensione dell'attività didattica in presenza, presenza, impedendo agli studenti di frequentare la comunità scolastica e di poter sviluppare quelle capacità sociali e relazionali che invece in questo disegno di legge vengono finalmente apprezzate, ha prodotto delle conseguenze drammatiche con cui facciamo ancora molto poco i conti. Anzi, tendiamo forse a sottovalutare il fenomeno e a non volercene prendere seriamente carico per affrontarlo. La scuola e i percorsi formativi hanno un obiettivo primario, ovviamente, che è quello della formazione degli studenti, ma nella formazione degli studenti un ruolo centrale lo giocano la socialità la capacità relazionale degli studenti. In questo senso, un altro elemento che va tenuto in considerazione e che mi auguro che venga sviluppato in queste linee guida di prossima formazione sono anche i NEET, cioè quei ragazzi nella fascia preadolescenziale e postadolescenziale tra i quindici e i diciannove anni che non frequentano né la scuola, né altri luoghi, cioè stanno chiusi in casa e non fanno nulla.

che vuol dire che c'è una grande domanda di socializzazione, di relazione, di comunità, di sviluppo di competenze non cognitive e trasversali, per valorizzare ciò che, in questo sistema scolastico così come è concepito,

su un noto quotidiano nazionale dice che l'Italia è prima nel mondo per la difficoltà denunciata dai suoi studenti di approcciarsi alla matematica, cioè gli studenti italiani sono in assoluto nel mondo quelli che hanno più difficoltà a studiare la matematica. È un dato che mi ha lasciato particolarmente sorpresa, e non tanto per la difficoltà nello studio della matematica, che forse chiunque abbia fatto gli studi classici come me in può anche condividere e comprendere, quanto perché pensavo che negli anni che sono trascorsi da quando mi sono diplomata fino ad oggi questa remora, questa difficoltà ad approcciarsi allo studio della matematica fosse superata e si fossero evoluti anche i sistemi didattici. Invece evidentemente non non è così. Quello che mi ha colpito molto di questa ricerca sulla difficoltà nello studio della matematica è il fatto che i sociologi che l'hanno redatta hanno evidenziato come il più grande fattore di stress e di impedimento all'acquisizione delle nozioni, e quindi della conoscenza della matematica, sia l'ansia: sancito proprio plasticamente che, quando si studia con l'ansia, non si riesce ad apprendere, i processi cognitivi si spengono, si annullano. Un disegno di legge come quello in esame sicuramente va incontro a questa necessità. L'unica cosa per la quale, francamente, come sempre, non posso che avere un moto di delusione nei confronti del Governo è la mancanza di risorse: anche il disegno di legge pur con tutta la sua buona volontà, le sue buone intenzioni, pur con tutta la capacità di prendere atto di un mutato quadro e di una necessità di adeguare la scuola ai nuovi contesti, poi tradisce le sue intenzioni e sacrifica anche le nostre aspettative; non disponendo di risorse specifiche, finisce per affidare come sempre tutto alla buona volontà del personale scolastico e al sacrificio dello stesso.

pedagogisti, cioè persone che possono dare un contributo per andare in questa direzione, lavorare in *équipe* e, quindi, in modo collettivo, sapendo

Signor Presidente, mi scuso già da adesso, ma parlerò per i miei dieci minuti. Oggi siamo chiamati ad affrontare un tema di straordinaria importanza qual è l'introduzione delle competenze non cognitive nei percorsi educativi. Pur riconoscendo le finalità nobili e condivisibili del disegno di legge, il testo, dopo un lungo *iter* che a far tempo dalla scorsa legislatura ne ha annacquato la portata innovativa, svilendone il valore, si presenta oggi alla stregua di un denaro finto che non compra, un mero elenco di buone intenzioni privo di concretezza e soprattutto di risorse adeguate. Le competenze non cognitive - come ognuno sa - comprendono abilità legate agli ambiti emotivi e psicosociali, dalle capacità comportamentali a tratti della personalità come l'apertura all'esperienza, l'estroversione, la creatività e la stabilità emotiva. Si tratta di competenze essenziali per formare individui non solo bravi studenti, ma anche cittadini responsabili, capaci di costruire relazioni e affrontare le difficoltà della vita. Tuttavia, mi chiedo come possiamo promuovere efficacemente tali competenze se non forniamo le risorse necessarie per farlo. Talvolta non è tanto importante innalzare un edificio, quanto vedere dinanzi a sé le fondamenta degli edifici possibili, ma non è questo il caso. Le scuole necessitano di programmi pragmatici, di formazione specifica per gli insegnanti e di un supporto finanziario con investimenti adeguati che permettano l'implementazione di tali progetti. Sicuri segni, i ripetuti, insistiti e più oscuri risvolti che quotidianamente ci riporta la pagina nera della cronaca ci dicono come le esperienze di disagio e vulnerabilità che i nostri giovani stanno vivendo richiedano un'attenzione affatto particolare da parte delle istituzioni. Tuttavia, il testo che stiamo esaminando non sembra farsi carico di questa urgenza, dacché, mentre discutiamo il disegno di legge sulle competenze non cognitive, ci corre l'obbligo di evidenziare una grave lacuna che permea questo provvedimento, ovvero la totale assenza di un *focus* sull'educazione emotiva, cioè sul creare uno spazio dove i giovani possano confrontarsi e sperimentare le loro esigenze. Si tratta di un aspetto cruciale che la maggioranza sembra ignorare. E non possiamo permettere che la nostra capacità educativa si limiti a un elenco di buone intenzioni, trascurando quell'ascolto volto a raccogliere le necessità fondamentali dei nostri giovani. L'educazione emotiva non è solo un complemento, ma è anche una necessità entro l'alveo di una società complessa e tale che le competenze non cognitive non possono essere dissociate da una solida formazione emotiva. Occorre avere una maggiore disponibilità di tempo da dedicare ai ragazzi. A tal proposito, sto lavorando a un disegno di legge specifico da affiancare agli altri dei colleghi concentrati sul tema, che prevede l'incremento del monte ore scolastico dedicato all'educazione emotiva, insieme all'istituzione di un fondo per l'aggiornamento degli insegnanti: una formazione continua fondamentale affinché i docenti siano adeguatamente preparati per determinare la formazione delle competenze emotive e sociali ai loro studenti. La mancanza di un *focus* sull'educazione emotiva nel disegno di legge in esame quest'oggi è pertanto una grave omissione, perché la vera educazione non può limitarsi a trasmettere conoscenze, ma deve anche creare le condizioni per coltivare il cuore e la mente. Come ha sottolineato Daniel Goleman, «l'analisi dell'analfabetismo emotivo è fondamentale per affrontare le sfide che i nostri giovani stanno vivendo oggi. Per questo motivo, è nostro dovere agire per prevenire forme di disagio che possono portare a comportamenti devianti, come il bullismo e il cyberbullismo. prosegue sostenendo che la capacità di riconoscere, comprendere e gestire le emozioni proprie e altrui è essenziale per il successo non solo in aula, ma nella vita. Immaginate un'aula dove i nostri ragazzi apprendono non solo la storia e la matematica, ma anche come comunicare in modo empatico, collaborare con i compagni e affrontare le sfide della vita attraverso la resilienza e una sana gestione del conflitto. Si tratta non di un sogno irraggiungibile, bensì di una possibilità concreta, ma ci vuole la volontà politica. Allo stesso modo, altri studiosi, come James Coleman, ci ricordano che le relazioni interpersonali sono fondamentali per l'apprendimento. In un'epoca segnata dalla solitudine, dall'isolamento e dall'indifferenza, dobbiamo ripensare le nostre scuole come comunità inclusive e accoglienti, in cui ogni studente si sente visto, ascoltato e valorizzato. È necessario rendere le scuole punti di riferimento per i cittadini, luoghi dove le famiglie si sentano supportate e aiutate a trovare risposte ai problemi che la vita ci pone. Le competenze non cognitive, come la capacità di formare legami significativi e di lavorare in *team*, devono diventare parte integrante del nostro vivere quotidiano. Dobbiamo fare in modo che ogni ragazzo possa privilegiare il potere del noi invece che subire il peso dell'io. Ribadisco, però, che tutto ciò necessita di un impegno concreto e sostenibile sotto il profilo economico: aspetti che sono totalmente assenti nel provvedimento

Infatti, nell'ambito di una sperimentazione nazionale, finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici, grazie al mio emendamento il Governo garantirà l'accessibilità di tali competenze anche agli studenti con disabilità e ai bisogni educativi speciali, promuovendo un'educazione realmente inclusiva ed equa. Tale proposta emendativa ci dà modo di ribadire come - a nostro giudizio - il sistema educativo non debba lasciare indietro nessuno, offrendo a tutti le stesse opportunità di apprendimento e sviluppo; una capacità di inclusione che non è solo una questione di equità, ma rappresenta anche un investimento che arricchisce l'intera comunità scolastica. Nel merito del provvedimento l'articolo 1 del disegno di legge reca disposizioni indirizzate a favorire e introdurre nei percorsi scolastici lo sviluppo delle competenze non cognitive. Come possiamo parlare, tuttavia, di successo formativo e di prevenzione della povertà educativa se non abbiamo una progettualità concreta per attuare queste idee? La teoria è ben scritta, ma manca pragmatismo. Le scuole necessitano di programmi concreti, di formazione adeguata per gli insegnanti, di spazi di socializzazione e convivialità, come ad esempio teatri, laboratori, cineforum, palestre e biblioteche. Serve quindi un investimento finanziario che permetta l'implementazione di questi progetti. Analogamente l'articolo 2 propone solo una mappatura di esperienze già esistenti, senza alcun piano concreto per integrarle nel *curriculum*. Dove sono le risorse destinate alla formazione degli insegnanti, alla creazione di programmi specifici e al monitoraggio dell'efficacia di queste iniziative? Soffermandoci poi sull'articolo 3, che prevede un piano straordinario di azioni formative per i docenti, mi chiedo che fine farà questa progettualità se mancano le risorse necessarie. L'articolo 4, infine, introduce una sperimentazione su scala nazionale, senza delineare però alcun vero e proprio percorso formativo. Onorevoli colleghi, in estrema sintesi, non possiamo permetterci di esprimere un voto favorevole su un disegno di legge che, sebbene apprezzabile nelle intenzioni, giunge sul filo di lana come un insieme di promesse vuote. È nostra responsabilità garantire che le politiche educative siano efficaci, concrete e sostenute da adeguate risorse. Sostenere lo sviluppo delle competenze non cognitive è essenziale, ma deve avvenire in un contesto di maggiore realismo e più ampia progettualità. Pertanto, il MoVimento 5 Stelle, convinto fermamente che i nostri giovani meritino più più di un semplice elenco di buone intenzioni, dichiara il suo voto di astensione sul provvedimento. Signor Presidente, la scuola, insieme alla famiglia, è il luogo deputato alla formazione dei giovani. Ciò significa che essa non può limitarsi a trasmettere il sapere, cioè istruire, ma deve anche educare, cioè impegnarsi affinché gli allievi possano sviluppare una loro personalità, forgiando forgiando il proprio carattere. Ciò è fondamentale per permettere loro di entrare in società da protagonisti attivi. Il compito dell'educatore, inoltre, è quello di tirare fuori da ogni individuo ciò che è già nel fondo della sua anima, che costituisce il suo essere, cioè la propria identità e personalità. La scuola ha svolto da sempre questo ruolo, ma negli ultimi decenni esso si è andato perdendo o assottigliando. Da qualche anno, però, anche nel mondo del lavoro si è cominciato a dare sempre più attenzione alle competenze non cognitive. Le *soft skills* o *life skills* sono richieste ai nuovi assunti per svolgere mansioni sempre meno meccaniche e sempre più creative. Non basta, infatti, sapere tante cose, ma occorre anche assumere in modo critico e creativo le nozioni che si sono apprese, integrandole nel proprio progetto di vita e facendole fruttare nella vita quotidiana. Più in generale, è la nostra società che ha sempre più bisogno di queste risorse, fra l'altro indispensabili per il buon funzionamento della democrazia. Si è infatti diffuso tra i giovani, negli ultimi tempi, un senso di insicurezza e disagio, che crea non pochi problemi, anche quando non sfocia - come purtroppo pure accade - in episodi di violenza. Si pensi solo al bullismo, all'aggressività diffusa, alla violenza contro gli insegnanti e agli altri studenti, oppure alla sempre più diffusa immaturità affettiva e all'incapacità di vivere i sentimenti e le emozioni senza lasciarsene sopraffare. Per non dire dello stress, il quale, non opportunamente gestito, può creare forti scompensi della personalità. Il lungo periodo del Covid-19 ha finito poi per accentuare, secondo molti studi, queste disfunzioni. Fra le conseguenze più vistose sono da considerare la mancanza di sicurezza e l'inefficacia manifestata nei rapporti interpersonali; la scarsa capacità di empatia, cioè della capacità di immedesimarsi nell'altro, e la scarsa consapevolezza di sé stessi e delle proprie capacità. Non poche volte si è poi incapaci di prendere una decisione di fronte a qualsiasi dilemma; incapaci, fra l'altro, di esercitare fino in fondo quei diritti che ci spettano in quanto cittadini. Per sviluppare tutte queste attitudini, considerata anche la complessità delle nostre società, la legge prevede opportunamente un'apposita formazione dei docenti che saranno preposti a questa attività. E la legge prevede anche una fase di sperimentazione, che inizierà già dal prossimo anno, propedeutica all'introduzione vera e propria delle attività di implementazione delle conoscenze non cognitive nei percorsi scolastici. Per tutto questo, consapevoli dell'importanza del progetto educativo che sta a monte delle disposizioni qui in esame, il Gruppo Lega dichiara il proprio voto favorevole al disegno di legge. tocca anche a me fare una piccola cronistoria, ma sarò molto rapida. Questo disegno di legge nasce nella scorsa legislatura: pressoché simile, ma aveva una cosa in più ed è l'unica cosa che qui manca e che ci costringe, nostro malgrado, ad astenerci. Nella scorsa legislatura avevamo trovato le risorse le risorse sono fondamentali per fare in modo che questo disegno di legge, che tocca un punto estremamente cruciale e serve alla scuola, possa davvero esplicare la sua efficacia.

abbiamo un disegno di legge che vedrà una terza lettura. Dopo essere partito dalla Camera, arrivato al Senato, qui la Commissione ha potuto apportare delle modifiche molto utili. E tornerà alla Camera con grande tranquillità, avendo consentito ai legislatori, per una volta, di svolgere bene il proprio lavoro. ringrazio sia il Presidente della Commissione, il presidente Marti, ma ringrazio anche il Governo, perché devo riconoscere che c'è stato uno scambio davvero attento e proficuo nell'elaborazione del percorso. Io voglio essere ottimista perché, essendoci un'altra lettura e sapendo che si sta lavorando per provare a costruire un fondo che possa dare respiro a questo disegno di legge, io mi auguro appunto che, nel corso della prossima lettura, possa esserci un appoggio complessivo e favorevole anche del Partito Democratico perché quelle risorse finalmente sono state ritrovate. Perché quelle risorse sono fondamentali, signor Presidente? Il Governo lo sa benissimo. Per rendere efficaci le competenze non cognitive e per non renderle una cosa a sé rispetto al percorso che si fa a scuola, unendole alle competenze cognitive, c'è bisogno di insegnanti formati. Alcune scuole sono già partite. Alcune scuole da anni portano avanti questo tipo di percorso e hanno messo in atto una didattica estremamente innovativa. Alcune di queste scuole, per esempio, sono quelle che hanno già sperimentato da anni, a partire dal 2014, percorsi quadriennali, perché avevano bisogno, dovendo modificare tutto il loro percorso di studi e facendo in modo di raggiungere gli stessi obiettivi in quattro anni, di modificare appunto la didattica, tanto che si parla di una didattica per competenze. Proprio in quest'Aula, quando abbiamo approvato i percorsi quadriennali e abbiamo abbiamo votato difformemente dalla richiesta del Governo, una delle motivazioni era anche questa: se anche in quei percorsi non aiutate i docenti a formarsi e a dotarsi di una didattica diversa e innovativa e ad essere pronti a rispondere a quelle esigenze, anche un obiettivo che può essere considerato positivo non viene raggiunto. È il tema delle risorse, Sottosegretaria, lei lo sa bene; un tema che, soprattutto quando riguarda la scuola, diventa fondamentale, perché noi non possiamo continuamente chiedere cose buone. Ripeto: questo disegno di legge disegno di legge tocca degli aspetti fondamentali. Non c'è un'opposizione che dice state sbagliando, perché lo sentiamo nostro. Come ha spiegato la collega Gelmini, l'abbiamo elaborato all'interno dell'intergruppo sulla sussidiarietà. È trasversale: ci sono forze politiche che si sono confrontate e hanno sposato il tentativo di portare avanti questa impostazione. Ma, se non abbiamo le risorse, anche quell'obiettivo diventa un'ulteriore fatica per le scuole, e paura. Una cosa che ci hanno detto molti mondi legati alla scuola, nelle audizioni, è stata quella di prestare attenzione, perché per come la state raccontando - e non è il vostro obiettivo - sembra che vogliate dedicare l'attenzione alle competenze non cognitive, dimenticandovi che, senza le competenze cognitive, il lavoro non riesce a farsi. E l'obiettivo non è questo, ma è invece proprio quello di lavorare insieme - lo provo a spiegare più semplicemente - e cioè lo svolgimento normale di un percorso di una disciplina, unito però alla modalità con cui sia il docente la insegna rispetto ai bisogni particolari che ha in quella classe; quindi in che modo riesce a modificare la classica lezione frontale per raccogliere le esigenze dei ragazzi che si trova davanti e cogliere, attraverso le loro emozioni, i loro bisogni e le loro sensazioni quegli apprendimenti che possono stare insieme. In che modo lo facciamo? Qui serve una didattica per competenze e la didattica per competenze la fai solo attraverso la formazione. In questo disegno di legge, togliendo qualsiasi possibilità, nonostante la buona volontà - devo dire - anche del relatore, che ha atteso fino all'ultimo nel tentativo di riuscire a trovare quelle risorse e quel fondo, si rischia di fare un po' un buco nell'acqua che noi vorremmo veramente evitare. Ripeto - e chiudo - che l'obiettivo è estremamente positivo, e per le nostre ragazze di crescere in un ambiente scolastico capace di interpretare i loro bisogni e, quindi, di parlare la loro lingua. Chi può non essere d'accordo? Ma, per fare questo, noi abbiamo bisogno di investire nel gruppo del consiglio di classe e del collegio docenti, offrendo offrendo loro gli strumenti affinché quella capacità didattica e quella nuova innovazione didattica possano essere davvero efficaci. Dobbiamo aiutarli a fare scuola, dando loro gli strumenti; il che vuol dire fare in modo di potenziare percorsi di aggiornamento e di formazione e, per fare quello, ci vogliono

che è attenta a questo aspetto, possano trovare quelle risorse che noi, con una serie di emendamenti trasversali, vi abbiamo chiesto. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Sottosegretario, il disegno di legge che oggi ci apprestiamo ad approvare parte da un assunto fondamentale: l'istruzione è un pilastro portante della società e che la scuola, oltre a formare le menti, forma le coscienze *(Applausi)*, e il progresso delle coscienze al progresso di una Nazione. Purtroppo viviamo tempi complessi, soprattutto dopo gli anni tragici della pandemia, che hanno messo a nudo tutta la nostra vulnerabilità, specie nei bambini e negli adolescenti. La scuola, oggi più che mai, è chiamata ad affrontare un'enorme sfida: quella di innovare l'azione didattica, anche e soprattutto con lo scopo di contrastare il problema dell'abbandono scolastico e dei giovani che non studiano, non lavorano e non si formano (i cosiddetti NEET). Solo obiettivi, questi, del PNRR, e quindi di primaria importanza per la nostra Nazione, che stiamo affrontando con grande impegno. Negli ultimi due anni, grazie al Governo Meloni e al ministro Valditara, si sono fatti passi in avanti. La dispersione scolastica - questo è un dato oggettivo

Questo risultato è stato raggiunto grazie a un lavoro mirato, a una serie di interventi messi in campo che hanno consentito di intervenire in maniera puntuale e non a chiacchiere, non a teorie, ma in pratica, con fatti concreti e inconfutabili, con Ha consentito di intervenire sul territorio e di coinvolgere i ragazzi sul piano didattico e sul piano delle competenze extracurriculari.

senso. È ormai assodato che il compito primario del percorso educativo e didattico non è la sola trasmissione dei saperi e l'acquisizione di competenze cognitive noi - Presidente, tramite la sua persona mi rivolgo alla collega Malpezzi - non dimentichiamo assolutamente; anzi, ribadiamo a gran voce che vogliamo le competenze cognitive. Ma l'istruzione deve riconoscere l'importanza dell'implementazione di tutte le competenze trasversali esistenti, comprese quelle non cognitive, per raggiungere obiettivi formativi Per questo oggi più che mai sono necessari percorsi scolastici che preparino le nuove generazioni ad avere abilità di gestione dello stress, apertura mentale, capacità di comunicazione, fiducia in sé stessi, negli altri, nella comunità; in poche parole, atteggiamenti positivi e corretti, con le giuste competenze, che rendano l'individuo capace di far fronte efficacemente alle richieste e alle sfide della vita quotidiana, anche nel campo lavorativo. Torno di nuovo a quei famosi NEET, di cui ho sentito parlare in diversi interventi. Questo è un punto su cui abbiamo fatto un intervento importantissimo:

ma noi, come scuola, non riusciamo a darle. Ecco che interviene il Ministero e fa questa grande riforma.

ha un obiettivo importante, che è quello di rendere gli studenti autonomi nel compiere delle scelte consapevoli

realmente cambiare il proprio futuro, in modo che si possa finalmente portare il ragazzo alla piena realizzazione della sua

I dati che anche in questi giorni sono stati presentati da Save the Children, ma anche dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, ci stanno dicendo come in Italia troppi bambini si trovino in povertà assoluta e tanti in povertà relativa. Sono percentuali da capogiro e che ci fanno dire che ci sono bambini che dormono in case non riscaldate, che non hanno un pasto proteico giornaliero, che non hanno i soldi per potersi comprare un libro, un libro, che non hanno la possibilità di svolgere una vita normale. E, quando non si svolge una vita normale in quella fascia d'età, si è a rischio e c'è il rischio che non si possano avere delle prospettive per il futuro. Quando parliamo dei diritti dell'infanzia, forse dovremmo parlare

che si occupano dell'infanzia e non le mette al centro della propria azione politica è un Paese che non investe sul futuro. Allora dico che in questa Giornata forse tutti noi dovremmo prendere l'impegno l'impegno di provare a realizzare, almeno da qui al prossimo anno, un grande intervento nei confronti dell'infanzia. Il primo tra tutti - ma ce ne possono essere altri potrebbe essere quello di avere finalmente una mappatura chiara sulla situazione degli asili nido e una possibilità importante di capire che fine ha fatto la garanzia infanzia: quel pacchetto di norme che sappiamo essere così importante *(Applausi)*, che proviene dall'Unione europea e che deve trovare deve trovare una condivisione per l'utilizzo, perché lì ci sono risposte che possono servire proprio a tutti i nostri bambini.

di povertà educativa, che spesso cogliamo in vari ambiti. È per questo che sono molto convinta del fatto che sia assolutamente fondamentale e rilevante che, per la tutela e la protezione dell'infanzia e dell'adolescenza, sia importante avere la massima compartecipazione possibile di tutte le forze politiche.

a trovare quella socialità che dovrebbe essere un elemento fondamentale del suo sviluppo, della sua evoluzione. Crediamo che questo sia un tema sul quale è bello e importante che vi sia massima compartecipazione. Per questo ho colto subito con entusiasmo la richiesta la richiesta della senatrice Malpezzi di fare questo momento di riflessione a fine seduta sul tema, perché sappiamo che su molte di queste tematiche vi è assoluta convergenza. Spero pertanto che potremo continuare a lavorare insieme per dare il nostro fattivo e concreto contributo, come vedo che il Governo sta facendo, per esempio, nel rinforzare i programmi scolastici per dare maggiore preparazione ai nostri ai nostri ragazzi, piuttosto che nel vietare l'utilizzo dello *smartphone* in classe perché - come dicevano i greci - il bene è nel mezzo. Noi andiamo quindi a valorizzare le tecnologie, ma dobbiamo anche salvaguardare la mente, lo sviluppo e l'evoluzione dei nostri bambini, perché vogliamo vogliamo crescere una gioventù libera e forte. in occasione del trentacinquesimo anniversario della approvazione, da parte dell'Assemblea delle Nazioni unite, della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata dall'Italia nel 1991, oggi si celebra la Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per sottolineare l'impegno a garantire loro l'opportunità di crescere e raggiungere il loro pieno potenziale. La Convenzione è uno dei trattati sui diritti umani più ratificata al mondo, ma - ahimè - è ancora ben lungi dall'essere attuata. Per esempio, la nostra stessa Italia

Oggi in Italia abbiamo ancora 1.295.000 minori che vivono in povertà assoluta (pari al 13,5% del totale), di cui 200.000 tra gli zero e i cinque anni (pari all'8,5 per cento del totale) che vivono in povertà alimentare, cioè non riescono a fare un pasto proteico ogni due giorni; in più abbiamo l'abbandono scolastico. Gli investimenti sono scarsi ed evidentemente insufficienti. Le politiche sono frammentate e inefficaci ed è vergognoso che quel che dovrebbe essere intollerabile si stia trasformando in accettabile. se passiamo a guardare quel che accade nel mondo, i dati sono drammatici e ci rappresentano che un miliardo di minori ogni anno è colpito da violenza, abusi fisici, sessuali, emotivi e abbandono, con conseguenze che rimarranno per tutto il resto della vita. I dati (si riferiscono al 2023) mostrano che un bambino su cinque (pari a 473 milioni) nel 2023 viveva in una zona di guerra; ogni giorno c'è stata una media di 31 bambini al giorno mutilati o uccisi; 17,6 milioni sono in uno stato di fame (questo dato è aumentato del 20 per cento rispetto a dieci anni fa). C'è anche il problema del cambiamento climatico: 300 milioni di bambini - quindi uno su otto - su scala globale hanno subito eventi meteorologici estremi con l'interruzione del percorso scolastico e dei percorsi formativi e 40 milioni di minori. Insomma, gli attivisti dell'infanzia di tutto il mondo si chiedono quali azioni compiere trovare la soluzione della crisi climatica, ma soprattutto per porre fine ai conflitti. Il nostro Paese dovrebbe impegnarsi per la promozione di soluzioni negoziali dei conflitti in corso, perché mi pare che l'età della clava sia abbastanza remota e dovrebbe essere subentrata quella della ragione. Ma, se continuiamo a investire in armi, in strumenti di distruzione e di morte, non so come faremo. Concludo facendo mie le parole del portavoce UNICEF James Elder: le grida dei bambini non si sentono, il silenzio del mondo diventa assordante e ancora permettiamo che l'immaginabile diventi il paesaggio dell'infanzia, una nuova normalità orribile e inaccettabile. vuole sensibilizzare tutti sul benessere di bambini, bambine e adolescenti, soprattutto nei contesti più difficili, e vuol riconoscere espressamente che anche i bambini, le bambine e gli adolescenti sono titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici che devono essere promossi e tutelati da parte di tutti. Condizioni di povertà, conflitti, violenze, cambiamenti climatici causano sofferenze a troppi bambini ancora oggi. Il compito degli adulti, quindi, e anche il nostro, dovrebbe essere quello di farli sorridere. Spesso ci domandiamo come riuscire a tutelare la loro dignità e il loro diritto a essere bambini, un periodo che dovrebbe essere fatto di gioco, di affetti, di momenti positivi; ad accompagnarli in un momento di crescita che dovrebbe essere sacro, poiché è in questa fase della vita che si costruiscono le basi di tutto quello che sarà l'adulto di domani. Purtroppo, ancora troppo spesso l'infanzia e l'adolescenza vengono negate o violate, anche attraverso matrimoni precoci o forzati, i cui numeri sono ancora impressionanti, o attraverso le mutilazioni genitali. promozione dei diritti umani del Senato assisteremo a un'audizione proprio su questo fenomeno, che riguarda 230 milioni di donne e ragazze che vi sono state sottoposte in giovane età e che sono segnate per sempre. L'audizione di domani riguarderà il fenomeno presente in Italia. Occorre, quindi, non voltarci dall'altra parte, occorre vigilare su tutti quei fenomeni che colpiscono i più piccoli e i più indifesi. La responsabilità di noi amministratori è quella di avere la massima attenzione nell'emanazione di provvedimenti che potrebbero avere ricadute anche involontarie sui bambini. Mi lasci, signor Presidente, esprimere un forte rammarico nell'apprendere dell'autorizzazione da parte del presidente Biden per la fornitura di mine antiuomo all'Ucraina. Sappiamo che proprio i bambini sono quelli più a rischio per questa tipologia di armi, motivo che portò alla sua messa al bando con il Trattato di Ottawa nel 1997. Spero che la notizia sia un *fake*, altrimenti sarebbe un triste ritorno al passato. vorrei sollecitare una risposta da parte del Ministro delle imprese e del *made in Italy* a una interrogazione che abbiamo presentato per conoscere quali siano le iniziative che il Governo, e in particolare il Ministro, intende assumere per assicurare una diffusione del servizio postale e degli altri servizi assicurati dalle Poste Italiane secondo criteri di prossimità Si moltiplicano, in questi giorni, le proteste e le lamentele da parte di molti cittadini nella città di Torino, che chiedono che non vengano chiusi diversi uffici postali che parrebbe invece Poste Italiane voglia chiudere. La questione merita una risposta e credo che il Ministro debba dare rassicurazioni e rispondere a tali richieste, che hanno - a nostro giudizio - un solido fondamento.